a causa di nostri errori ed incertezze - l'aggettivo nostri è riferito alle forze del centrosinistra e ai riformisti oggi raccolti nel Partito Democratico - la maggioranza dei cittadini italiani è convinta che in tema di federalismo fiscale le cose negli ultimi anni siano andate più o meno così: uno schieramento, il centrodestra, egemonizzato sul tema del federalismo dalla Lega Nord che preme per la svolta federalista, e uno schieramento, il centrosinistra, egemonizzato dalla sinistra statalista e centralista che resiste a questa innovazione temendo per l'unità nazionale. la semplice e banale cronaca di questi anni racconta una storia, secondo me, del tutto diversa. Rapidamente riassumo i passaggi essenziali di questa storia. il federalismo fiscale entra nella Costituzione per iniziativa del centrosinistra, che per introdurlo nel nostro ordinamento costituzionale compie un'inaudita forzatura politica: riforma della Costituzione a stretta maggioranza e autoproclamazione del successivo *referendum* che conferma l'innovazione introdotta.

I cinque anni passano, ma l'articolo 119 rimane totalmente inattuato. Perché il centrodestra voleva di più - come si è detto - con la riforma della devoluzione?

l'articolo 119, è possibile concludere che il centrodestra quell'articolo 119, così come era scritto e così come resta scritto in Costituzione, lo condividesse. Se lo condivideva - torna la domanda - perché in cinque anni di Governo, con tranquilla e straripante maggioranza, quell'articolo non è stato attuato? La risposta è semplice: perché nel centrodestra, in tema di federalismo fiscale, hanno avuto la prevalenza nel passato più o meno recente le forze ostili alla riforma, l'esatto opposto di ciò che racconta la vulgata massmediatica a proposito di federalismo fiscale. Nel centrosinistra prevale con fatica una posizione favorevole; nel centrodestra prevale con fatica una posizione contraria. La prova di tutto ciò è offerta dai 15 stentati mesi del Governo Prodi (terzo passaggio fondamentale). Il Consiglio dei ministri, infatti, approva un disegno di legge delega per l'attuazione dell'articolo 119, cioè il Consiglio dei ministri del Governo Prodi fa quello che il Governo precedente non era riuscito a fare: approvare un disegno di legge in Consiglio dei ministri in ben 60 mesi di attività. Il disegno di legge delega è approvato in Consiglio dei ministri dal Governo Prodi (ripeto, ciò che il Governo di centrodestra in 60 mesi non era riuscito a fare)

di attuazione dell'articolo 119, forse per farsi perdonare i cinque anni di totale inattività che erano appena trascorsi, ossia il disegno di legge della Regione Lombardia; quello è il riferimento preciso, puntuale del programma elettorale del Popolo della Libertà, un disegno di legge fondato su una interpretazione rigidissima del principio di territorialità delle grandi imposte erariali e sulla perequazione orizzontale tra Regioni. Il Partito Democratico, nel corso della campagna elettorale, presenta invece un programma che è incentrato, a proposito di federalismo fiscale, su una vera e propria autonomia impositiva del sistema delle autonomie locali, perequazione verticale e non orizzontale, fabbisogni ottimali standard, in termini di qualità e quantità, dei fondamentali servizi ai cittadini a cui uniformare le annuali decisioni

e molto propagandate naturalmente, ma solo tracce, dei due principi cardine del disegno di legge della Regione Lombardia, che per il resto viene abbandonato: territorialità di tutte le grandi imposte erariali e perequazione orizzontale. Nel disegno di legge Calderoli restano le tracce di quell'ispirazione, solo le tracce. Noi del Partito Democratico abbiamo tenuto in Commissione e terremo ora in Aula l'atteggiamento proprio della forza che ha dato il maggiore contributo; lo si voglia riconoscere o meno, questi fatti (io ho citato dei fatti di cronaca, non delle interpretazioni; fatti di cronaca, tempi, iniziative, approvazioni in Consiglio dei ministri, proposte presentate o non presentate, attuazione di articoli costituzionali o non attuazione) attuazione) dimostrano che la nostra è la forza che ha dato il maggiore contributo alla riforma federalista in Italia. Quindi, non abbiamo presentato singoli emendamenti

non sarebbe stata coerente con l'insieme dell'iniziativa sviluppata negli anni dai riformisti del centrosinistra. Abbiamo pertanto presentato un nostro disegno di legge organico, dal quale abbiamo fatto derivare le proposte emendative al testo Calderoli. Si è trattato di un'iniziativa seria ed efficace. Il testo approvato in Commissione dalla maggioranza, con il nostro voto di astensione, è stato profondamente influenzato dalle nostre proposte, e credo che questo sia giusto riconoscerlo, sia da parte nostra che da parte del Governo e della maggioranza. Restano aperte rilevanti questioni di merito, già riassunte brillantemente dal relatore di minoranza, senatore Vitali, che adesso non riprendo. Voglio solo richiamarne una. A mio avviso, può e deve essere meglio chiarito che il federalismo fiscale a regime, dopo la fase di transizione, dovrà assumere a base della legge annuale di stabilità della finanza della finanza pubblica un piano di convergenza che assuma e aggiorni sistematicamente gli obiettivi di fabbisogno ottimale standard per quantità e qualità dei servizi essenziali da fornire ai cittadini. modo verrà garantita la capacità del sistema di perseguire dinamicamente il riequilibrio nella quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini nelle diverse parti del territorio nazionale, escludendo cioè un'interpretazione del federalismo fiscale fondato su costi e fabbisogni standard che si limiti a fotografare l'attuale situazione che, come ben sappiamo, in termini di fornitura dei servizi ai cittadini italiani è fortemente sperequata tra le diverse Regioni italiane, e non sempre e non solo per responsabilità di cattivo governo da

per arrivare fin qui, sentiamo la responsabilità di costringere la maggioranza a condividere l'urgenza di un intervento riformatore che introduca, da subito, contestualmente all'approvazione di questa legge delega - naturalmente parlo di contestualità politica - il Senato federale. Nulla di ciò che possiamo ora decidere potrà essere attuato e gestito con efficacia e coerenza, portando responsabilità e trasparenza dove oggi regnano scaricabarile e opacità, senza una vera Camera delle Regioni liberata dal vincolo del voto di fiducia e del sostegno al Governo; nulla, compresa la sede di analisi tecnica dei dati di finanza pubblica. Senza la creazione di un vero *Congressional un Servizio del bilancio del Parlamento italiano, articolato in Camera politica e Camera delle Regioni, non si supera la logica opaca e consociativa cui siamo oggi costretti a tener dietro e sarà sempre dietro l'angolo il rischio che una delle parti in causa (Regioni, Stato centrale) blocchi il processo, contestando la parzialità del fornitore e dell'elaboratore dei dati di finanza pubblica posti a base delle scelte del decisore politico. Non si tratta, come risulta evidente dal lavoro svolto fin qui, per quel che riguarda

tratta di una posizione volta a motivare il disimpegno politico, al contrario. Si tratta di uno sforzo volto a garantire che l'impegno di oggi possa davvero essere fruttuoso arrivando alla piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Cosa chiediamo al Governo e alla maggioranza, signor Ministro? È semplice: di inscrivere subito all'ordine del giorno dell'attività parlamentare il disegno di legge di riforma del Parlamento elaborato consensualmente nella Commissione affari costituzionali della Camera alla fine della scorsa legislatura. Se avremo la Camera delle Regioni già

avremo creato le condizioni per attuare davvero l'articolo 119 della Costituzione. Non sarà stata una manovra propagandistica, né da parte vostra né da parte nostra, ma la premessa di un vero, radicale cambiamento della pubblica amministrazione italiana e con essa dell'intero Paese.

oggi è veramente un grande giorno. Si potrebbe definire una giornata veramente solare: stiamo scrivendo una nuova ed importante pagina della nostra storia, meglio ancora sarebbe dire un vero capitolo. Stiamo dando un futuro, certezza e sicurezza a milioni di famiglie ma, ancor di più, stiamo dando serenità e fiducia a milioni di giovani che si stanno affacciando alla vita sociale. Con questo atto e legge fondamentale la Lega rispetta in soli nove mesi il patto con i propri elettori. È come un bambino che noi cureremo e faremo crescere e non abbandoneremo mai. Ma la Lega dice anche grazie a tutto il Nord, con i suoi milioni di abitanti, che così gestiranno direttamente le proprie risorse per svilupparsi e progredire. Ed alla Lega dice anche grazie tutto il Paese, che così ora avrà la possibilità di dimostrare che le intelligenze, le capacità e le volontà esistono nell'area alpina come in quella mediterranea (non mi piace la contraddizione che spesso sento dire di Sud verso Nord) e si affrancherà così da un assistenzialismo che frena lo sviluppo e mortifica le coscienze. Non si dica che il federalismo divide il territorio, anzi, è proprio vero il contrario: federalismo, infatti, significa un patto tra comunità, tra genti, che parte dal basso e non è certo lotta e disaccordo. Chi in questi anni ha bloccato la riforma con bugie e disinformazioni, com'è anche avvenuto con i *referendum* sulla *devolution*, ha solo cercato di difendere posizioni personali di potere a danno dei cittadini; ma la verità emerge e ormai è un'onda impetuosa che non si può più fermare. Invero, è proprio ora che il Paese è diviso e questo non è più tollerabile e tollerato dalla nostra gente;

Si vede benissimo che se tutto il Paese applicasse gli standard e la spesa del Veneto e della Lombardia già ora avremmo ogni anno circa 3 miliardi di euro di risparmi e di minore spesa a parità di servizi e di qualità, che sarebbero anzi tra i più eccelsi, essendo riconosciuta

fossero rapportate agli enti più virtuosi o a quelli che usano in maniera oculata il denaro pubblico, come ad esempio le città di Torino, di Venezia, di Bolzano o di Trento, ogni anno ci sarebbe sicuramente almeno un miliardo di euro di minori costi e certamente i servizi resi ai cittadini non scadrebbero di qualità; anzi, sarebbero forse di qualità È giusto ricordare alcuni dati, perché spesso abbiamo sentito nelle discussioni che forse certi dati di paragone per quanto riguarda le novità che porterà il federalismo fiscale non esistono. I dati li conosciamo bene e vorrei appunto qui riprenderli.

interessante anche vedere il dato sulle contravvenzioni *pro capite* nel nostro Paese: Napoli è uguale a Torino con circa 77 euro *pro capite*, ma credo che gli effetti dei servizi nelle due città siano davanti agli occhi di tutti.

diversità di trattamento o a parità di entrate ma con diversità di gestione dei servizi, è abbastanza evidente. Interessante è anche studiare la spesa *pro capite*. Tra le prime città in Italia vediamo ancora Napoli, spende 1.500 euro per abitante di sola spesa corrente, con un valore praticamente pari alla media esistente tra le spese correnti e d'investimento di tutte le maggiori città. Ovviamente, ciò sta a significare che vi è un fortissimo il totale della spesa di Napoli è di circa 2.300 euro per abitante: esattamente il doppio di una città come Novara che spende soltanto 1.165 euro

Se poi guardiamo allo stato delle priorità per macro Regioni in Italia, vediamo che al Nord prevalgono le spese nell'istruzione, nella cultura e nel settore sociale;

Veniamo ora al discorso delle spese di autoamministrazione, perché queste sono abbastanza emblematiche. Quali sono le prime sei città in Italia in

Bari, Trento, Bolzano, Roma, Torino e Venezia, chiaramente in ordine decrescente dal 23 per cento di Bari al 20 per cento di Venezia. Ovviamente, noi non pensiamo che in tutta l'area mediterranea manchi la capacità di spendere in maniera oculata. Vi sono esempi che possono essere presi in considerazione, ma la tendenza è quella che prima evidenziavo. In effetti, questi studi dimostrano che la spesa corrente, mediamente, nelle realtà mediterranee si attesta tra il 30 e il 31 per cento con incrementi di spesa corrente annua, sul 2007 rispetto al 2006, tra l'8 e il 9 Grazie. che con questo federalismo riporteremo in equilibrio il Paese e daremo la possibilità a tutte le realtà di confrontarsi su parità Grazie.

Grazie.

Devo e voglio esprimere un fortissimo ringraziamento ai ministri Bossi e Calderoli per il grande ed impegnativo lavoro svolto: a loro va un caloroso abbraccio. A Bossi rivolgo un grande applauso per aver sempre guidato e per guidare ancora con coraggio, determinazione, lucidità e lungimiranza la Lega Nord, sventolando e tenendo alta la bandiera del federalismo. Non dimentichiamo che la Lega Nord è un movimento federalista, un'unione feconda di tanti movimenti ed io parlo per il grande e nobile popolo veneto, come Lega Veneta. Il nostro riferimento veneto è San Marco, come sintesi delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Benissimo ha fatto poi il ministro Calderoli a partire dal basso, dalle istituzioni vicine alla gente, dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni, nella formulazione del provvedimento; non poteva comunque fare diversamente perché così si costruisce il vero federalismo.

Tutte le parti politiche hanno riconosciuto che un lavoro così profondo, approfondito, appassionato e produttivo non si vedeva da molte legislature. un riconoscimento sincero al relatore Azzollini per lo sforzo prodotto, così come desidero citare il presidente e coordinatore Baldassarri per le mediazioni e l'equilibrio nei lavori. Rivolgendomi all'opposizione mi sarebbe facile sottolineare che, dopo neanche un anno, siamo arrivati all'obiettivo, mentre loro in due anni, nella passata legislatura, non hanno cavato poco più o poco meno di un ragno dal buco.

Non siamo per il muro contro muro. Invito, dunque, a rompere i vecchi schemi e a dimostrare coraggio politico, esprimendo un voto favorevole e dando un segno tangibile al Paese che la classe politica è cambiata.

di essere uguale al Paese e di sapere esprimere in maniera forte un sì convinto. Sterili polemiche e ricattini che ho sentito anche in quest'Aula, ma che non hanno senso, abbandoniamoli. Termino: ora siamo come dei Padri costituenti e dobbiamo dare unitamente futuro e certezza al Paese, una testimonianza speciale di speranza. Grazie.

l'Atto Senato n. 1117, disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, ha lo scopo di dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, così come modificato dalla riforma del Titolo V della Parte II, introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel quadro della ridefinizione dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali anche in materia tributaria e, più in generale, nel settore della finanza pubblica. Si tratta sia di un atto dovuto, come la Corte costituzionale ha ripetutamente evidenziato, che di una grande opportunità per il Paese, per mettere in moto un processo virtuoso tale da portare ad una maggiore efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione nel suo complesso, ma anche della responsabilità degli amministratori. Tuttavia, un'attuazione distorta e strumentale può mettere in pericolo l'unità del Paese e i diritti dei cittadini, in presenza di un quadro istituzionale ancora indefinito riguardo alla distribuzione delle funzioni tra i livelli di governo e, in conseguenza, di grandezze finanziarie non ancora quantificate né quantificabili. II punto qualificante della riforma, ovvero il passaggio dal criterio della cosiddetta spesa storica - fondato sul sistema dei trasferimenti statali effettuati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti - a quello dei cosiddetti costi standard, relativi all'individuazione di una misura uguale in tutto il territorio nazionale per l'erogazione delle prestazioni (al netto quindi delle inefficienze e degli oneri aggiuntivi), è il vero nodo, che non è stato ancora sciolto in maniera sufficiente. Quali saranno le modalità e i criteri guida nella determinazione dei costi standard? Tale operazione è assai complessa, in quanto i criteri per determinare i valori standard non possono riguardare solo i costi efficienti, ma devono coinvolgere anche l'omogeneizzazione della quantità di servizi e di dotazioni infrastrutturali, e non può essere rimessa per intero al Governo con l'ausilio della Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4. Sembra assente, nel disegno di legge in discussione, la trasparenza quanto ai dati finanziari, che soli possono illuminare sulle reali conseguenze del disegno di legge Qui ci sono due elementi da richiamare: innanzitutto, è difficile disporre nel nostro ordinamento di dati affidabili senza una previa riforma della contabilità di Stato e di quella regionale, che seguono ad oggi sistemi diversi. Inoltre, si tratta di dati di cui comunque dispone il Governo, a cui fanno capo la Ragioneria generale dello Stato e l'ISTAT. Essi dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento, che dovrebbe poterli verificare tramite il suo Servizio di bilancio. Si tratta di un aspetto di genericità della delega, che viene esercitata in assenza di qualsiasi riferimento a dati concreti, che sarà possibile solo nel momento dell'adozione dei decreti legislativi; ma, a quel punto, il Parlamento si sarà già spogliato della sua potestà legislativa. II disegno di legge sembra abbia anticipato il necessario scioglimento di una serie di nodi ancora aperti nel Titolo V, che non a caso sono affrontati soltanto nelle disposizioni transitorie,

la specificazione del termine da cui decorre il periodo medesimo. L'Italia dei Valori ha sempre dimostrato condivisione su un federalismo fiscale solidale, che introduca una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli amministratori e degli enti locali. Ma la concreta azione politica del Governo si pone in contrasto con l'intento dichiarato di riformare il sistema della finanza pubblica in senso federale; è il caso, ad esempio, dell'abolizione dell'ICI, che ha privato i Comuni di un importante strumento di autonomia tributaria, del finanziamento all'Alitalia e, più recentemente, del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Atto Senato n. 1195). L'articolo 16, comma 19, di tale provvedimento, infatti, ha la finalità di privare gli enti locali della titolarità di fondamentali compiti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, in contrasto anche con il riparto delle competenze amministrative previsto dalla Costituzione. Si assiste, infatti, all'estromissione delle amministrazioni regionali dalle procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione agli interventi di sfruttamento

Anche le decisioni assunte negli ultimi tempi dal Governo, che hanno visto un indiscriminato apporto di risorse alle amministrazioni regionali e comunali in difficoltà finanziarie, contraddicono l'obiettivo di un federalismo fiscale responsabile favorendo, al contrario, gli enti con una gestione inefficiente e non trasparente delle risorse pubbliche. Si potrebbe anche condividere il superamento del criterio della spesa storica, a patto di una maggiore definizione del fabbisogno standard al quale è attribuito il compito di razionalizzare e riqualificare la spesa delle autonomie territoriali. In tale settore occorre infatti considerare che anche negli ordinamenti di carattere più spiccatamente federale si procede alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni a garanzia dei cittadini, ma non necessariamente all'individuazione di un costo uniforme di produzione del servizio. L'autonomia finanziaria che si intende realizzare potrebbe comportare forti squilibri nella ripartizione delle risorse, anche favorendo alcune Regioni, con il pericolo di un incremento della pressione fiscale generale, oppure di una diminuzione dei livelli dei servizi essenziali, in tal modo vanificando la funzione assegnata al fondo perequativo. Emerge, dunque, il rischio che si assuma a parametro di riferimento la media delle spese sostenute da una singola Regione per uniformare i livelli standard in tutte le altre non tenendo conto delle differenti dotazioni di servizi e infrastrutture nelle varie parti del Paese. Il decentramento finanziario e fiscale che il Governo intende porre in essere se da un lato assume a parametro il fabbisogno medio delle Regioni e degli enti locali, dall'altro, tuttavia, non si preoccupa di delineare in maniera sufficientemente approfondita la natura e le caratteristiche delle funzioni demandate ai singoli livelli di governo prospettando inoltre anche una certa complicazione nella struttura contabile del fondo perequativo per i Comuni e le Province che si fonda sulla creazione di due conti distinti all'interno del bilancio regionale. Tale incertezza sussiste anche dal lato delle entrate degli enti decentrati le quali sono limitate, nel testo in esame, all'attribuzione di una riserva d'aliquota sulle basi imponibili di tributi erariali e sulla devoluzione del gettito di imposte statali per far fronte al trasferimento di competenze. Occorre, quindi, definire meglio le caratteristiche fiscali della riserva d'aliquota riconosciuta alle Regioni, soprattutto in riferimento alla disciplina dell'IRPEF. Infatti, il disegno di legge presentato dal Governo avrebbe dovuto chiarire quali quote del gettito dell'IRPEF si intendono attribuire alle Regioni per finanziare le loro funzioni fondamentali, considerando anche che tale gettito sembrerebbe destinato a disperdersi tra i vari enti subregionali. Emerge, dunque, un quadro particolarmente complicato e contraddittorio che sarebbe possibile razionalizzare facendo ricorso al modello fiscale di altri ordinamenti.

Chi pagherà questo debito pubblico? Chi pagherà l'esposizione dei Comuni, ossia circa 40 miliardi di euro di prodotti derivati? Queste sono solo alcune questioni.

Sono presenti ai nostri lavori, in occasione della loro visita al Senato, studenti dell'Istituto tecnico-industriale "Enrico Mattei" di Eboli. A loro e ai loro insegnanti rivolgo un saluto e gli auguri per i loro studi.

incontri, dibattiti, convegni, conferenze unificate, commissioni, e chi più ne ha più ne metta. Penso che ci sia stato il tempo necessario per discutere con calma di

quella federale dello Stato. Siamo di fronte ad una svolta; siamo all'approdo di quel federalismo fiscale per il quale la Lega Nord si è battuta con tenacia e coerenza - e credo che nessuno possa negare questo - convinta, ieri come oggi, che sia l'unica chiave in grado di scardinare il sistema centralista ed aprire la strada per la piena affermazione delle autonomie locali. Abbiamo celebrato lo scorso anno il 60° anniversario dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, ed è il caso di ricordare come proprio il tema delle autonomie (tema cardine della Costituzione della nostra Repubblica) non sia stato svolto nella pienezza delle sue aspirazioni e potenzialità. Non dimentichiamo che le Regioni sono state attuate nel 1970 e che, prima di acquisire pienezza legislativa, sono passati molti anni. Se pensiamo poi ai Comuni e alle Province, dobbiamo ricordare che fino a pochi anni fa ci siamo mossi nel tracciato del Testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, e mi pare che la data sia eloquente.

ma si è trascurata, quando non disconosciuta, la questione delle risorse, che non hanno avuto quell'incremento che facesse tornare l'equazione tra una domanda sociale sempre più articolata ed una risposta spesso condizionata da bilanci e da patti più o meno stabili. Basta ascoltare i sindaci, e gli amministratori in genere, per capire che occorre cambiare rotta in modo strutturale, e non trasformando gli amministratori in ragionieri di complemento. se fanno i *travet*, le mezze maniche, non vanno oltre la modesta ed ordinaria amministrazione; se ci mettono un po' di fantasia rischiano il giudizio della Corte dei conti e magari il danno erariale,

da questa fase dialettica e mettere in azione tutti i meccanismi che possano restituire ai territori le risorse che producono e che meritano, in modo che sia esaltato - lo abbiamo sentito ripetere molte volte in quest'Aula - il concetto di responsabilità e vengano premiate le amministrazioni virtuose. Le voragini aperte in alcune Regioni e Comuni hanno il potere di scoraggiare chi è attento ai bilanci e non vuole lasciare eredità passive e debiti ai loro successori e quindi ai cittadini.

esprime. Colleghi senatori, questa spirale di irresponsabilità morale e politica è la stessa che ha portato a livelli catastrofici e immorali il debito pubblico - l'ha ricordato il senatore Lannutti - in ragione del quale scandalosamente ciascun italiano nasce indebitato. Quindi, il federalismo fiscale è l'unica via o almeno una delle vie principali per ridefinire una strategia di valori e un impianto di strumenti e procedure che ridia fiducia, responsabilità ed autonomia. Non è secondario che il federalismo fiscale venga varato in una situazione finanziaria ed economica così preoccupante. Al contrario di chi ritiene che questo federalismo moltiplichi gli effetti debitori,

è l'unico antidoto ad una deriva che renderebbe il nostro Paese fanalino di coda, come è accaduto quando l'Italia è stata retrocessa al quarantesimo posto, dopo la Thailandia e la Lettonia, sul piano della competitività.

il frutto di risparmi - e spesso l'unico bene che umili famiglie lasciano in eredità ai figli - e in secondo luogo che si vuole agire con imposte inique per il mancato trasferimento di finanziamenti dal potere centrale a quello locale. locale. Nella proposta federalista sono contenuti tutti gli equilibri perequativi e solidali per togliere fondamento all'alibi di

ora è diventata indispensabile per la stessa tenuta dello Stato nelle sue articolazioni istituzionali dettate dalla Costituzione.

dal Battista, viene indicato proprio come l'Agnello di Dio. Due discepoli di Giovanni il Battista, a quel punto, seguono il Cristo, il rabbì (che

che gli amici della Lega insistono nel definire federalismo, ma che noi che siamo autonomisti per memoria (da molto prima che nascesse il federalismo)

sosteneva che le istituzioni (e quindi anche le leggi) fossero il vestito della realtà. Non possiamo pensare che la legge sostituisca o alteri la realtà. Ebbene, questo disegno di legge è una gigantesca e

recita testualmente: «Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome». Non è autonomo il Comune come ente o la Regione come istituzione, ma sono autonome prima È vero, quindi, che dobbiamo sforzarci come legislatori di costruire l'intelaiatura che serve a proteggere questa autonomia, ma penso che siamo andati oltre nel costruire un sistema fatto di tante deleghe, per noi parlamentari - oggi di opposizione, ma ambiamo a diventare forza di Governo (quindi vale oggi per noi e può valere domani per i colleghi dell'attuale maggioranza)

A me va bene che si dica - come ha fatto poco fa il collega della Lega - che si forza la mano quando si afferma che l'ICI sulla prima casa

Andrò al dunque dicendo una cosa anche al senatore Pastore, il quale stamane credo abbia commesso - non me ne voglia - un errore di entusiasmo

- dice testualmente il senatore Pastore - perché l'organo regionale «è il punto di riferimento del federalismo fiscale». Questo è un errore perché la nostra Costituzione ha stabilito una cosa che i federalisti di tutto il mondo capiscono quando la leggono: il nostro, se lo è, è un sistema federale molto particolare fondato sulla cosiddetta equiordinazione, termine complicato ma molto ben comprensibile. Se dunque noi a livello di Costituzione abbiamo questo principio saldo ma poi organizziamo un sistema con questa delega e la maggioranza, attraverso il senatore Pastore, dice che la Regione è l'organo di riferimento, è chiaro che stiamo facendo una cosa sbagliata. concludo dicendo che se ci sporgessimo un po' al di là di tutto quello che è scritto in questo complicatissimo disegno di legge e ci sforzassimo di capire che il problema non è individuare qual è il costo dell'asilo nido nell'ultimo paese della Calabria - senza dubbio sarà anche quello il problema - ma il problema - ma registrare che sulle grandi voci di spesa dello Stato e della Repubblica italiana (la previdenza, la sanità e l'assistenza) vi è un'eccedenza di spesa. Ciò è vero, ma è concentrato nelle Regioni più ricche: il prodotto interno della Lombardia, fatte le debite proporzioni, non è in linea con la spesa previdenziale della stessa Regione Lombardia e via dicendo. Allora, noi facciamo bene a compiere questa operazione che ha l'obiettivo di avvicinare il centro di spesa alla responsabilità di chi determina la spesa. Lo abbiamo fatto già in passato, però non credo che con questo provvedimento noi raggiungiamo l'obiettivo e non credo che questa sia la vera rivoluzione di cui si vuole parlare.

la Costituzione del 1948 ha dentro di sé un grande spirito autonomista. Lo ha detto il ministro Tremonti; è nei verbali delle nostre Commissioni. Vorrei finire proprio così:

in termini astratti e generali, noi - in questo caso mi faccio carico delle generazioni precedenti che hanno calcato la scena politica - avremmo esercitato ed immaginato un sistema centralistico dove Roma è ladrona e dove tutto viene sequestrato dal centro? Mi pare che ideologicamente c'è solo qualcuno che ha esercitato una forzatura e, forse, ancora oggi la vuole esercitare. *(Applausi Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo finalmente giunti alla discussione e all'approvazione del disegno di legge sul federalismo fiscale. Utilizzo, non a caso, la parola finalmente. Il federalismo fiscale arriva, infatti, in quest'Aula con oltre 7 anni di ritardo. Tanti ne sono trascorsi da quando il Parlamento approvò la riforma del Titolo V della Costituzione, poi ratificata dal popolo italiano il 7 ottobre dello stesso anno con il *referendum* confermativo. Nel 2001 il Governo di centrodestra invece di riprendere la modifica costituzionale approvata dalla maggioranza di centrosinistra preferì accantonarla per cimentarsi in un'ulteriore riforma chiamata *devolution*. Seguirono 5 anni impiegati per produrre l'ennesimo testo costituzionale che poi è stato bocciato dai cittadini con il *referendum* del 25 e 26 giugno 2006. Se nel 2001 fosse stato adottato subito il federalismo fiscale, peraltro in una congiuntura economica certamente più favorevole di quella attuale, oggi potremmo già apprezzarne gli aspetti positivi. Invece, quella che discutiamo in queste ore, nel bel mezzo di una gravissima crisi economica e sociale, è una riforma portata in Parlamento senza che vi sia stata la previsione di alcun tipo di risorsa aggiuntiva. Anzi, il testo non contiene neanche l'ombra di un numero o di un'aliquota. E, badate bene, stiamo parlando di materia fiscale! Spero poi che nessuno si sorprenda del fatto che, per attuare il federalismo fiscale, saranno necessarie maggiori risorse. Sul punto vorrei richiamare l'attenzione dei più distratti tra noi: per riuscire ad attuare il federalismo fiscale sarà necessario garantire alle diverse istituzioni, a tutti i livelli, le stesse risorse di cui hanno beneficiato finora, mentre i territori che oggi sono penalizzati, con un rapporto squilibrato fra le entrate tributarie prodotte e le risorse trasferite, dovranno ottenere fondi aggiuntivi. Il risultato è chiaro: nel complesso il federalismo fiscale ci costerà molto di più, quantomeno nella fase di avvio. Non potete negarlo, per far partire il federalismo nei primi cinque anni servono più risorse; poi gli effetti della riforma sull'efficienza e sulla lotta all'evasione inizieranno a dare i loro frutti. i 4 miliardi di euro che avete buttato per le vostre sciagurate scelte su Alitalia oggi sarebbero stati utilissimi per avviare questa riforma. Quando il centrosinistra approvò, nel 2001, la riforma del Titolo V, la spinta principale veniva dalla constatazione dell'anomalo funzionamento dei diversi livelli istituzionali e dell'iniqua distribuzione delle risorse nel Paese. Nonostante alcuni spunti importanti, l'attuazione della riforma è rimasta incompleta. Permane una confusione di ruoli fra le diverse realtà amministrative, con frequenti accavallamenti delle responsabilità fra Stato, Regioni, Province e Comuni. La conseguenza è che i cittadini e le imprese, che hanno la necessità di interloquire con la pubblica amministrazione, si trovano contro un impenetrabile muro di gomma che li fa rimbalzare tra i diversi uffici interessati; un inestricabile labirinto di competenze, di norme, di cavilli. L'esigenza di semplificare è, dunque, più viva che mai. Il Partito Democratico ha proposto, fin dall'inizio, che nel testo confluissero anche le norme sul funzionamento delle autonomie locali (la famosa Carta delle autonomie). Purtroppo non siamo stati ascoltati e le regole fondamentali su "chi fa cosa" fra i diversi livelli istituzionali non ci sono. Questa mancanza si tradurrà in una grande difficoltà nello stabilire i vari costi standard dei servizi per stabilire il giusto fabbisogno di ogni territorio. Creare una pubblica amministrazione più efficiente è uno dei due obiettivi prioritari della riforma federale. L'altro è rendere più equa ed equilibrata la distribuzione e l'utilizzo delle risorse, che la pubblica amministrazione nel suo complesso raccoglie ed eroga. Avvicinare il luogo in cui viene effettuato il prelievo fiscale a quello in cui le stesse risorse vengono impiegate per realizzare opere o per dare servizi incentiva il senso civico dei cittadini e aumenta la loro sensibilità nella lotta all'evasione fiscale e agli sprechi. Certo, per incentivare il senso civico servono norme fiscali semplici e chiare. Solo così il cittadino riesce a comprendere dove vanno a finire le tasse pagate. Nelle Regioni a Statuto speciale, ad esempio, i cittadini sanno già oggi quanto resta nel territorio. Purtroppo, la riforma che stiamo discutendo e votando non contiene questa semplificazione. Non chiarisce, inoltre, in che modo si intende affrontare lo squilibrio esistente fra le risorse assegnate alle Regioni a Statuto speciale rispetto a quelle ordinarie. Proprio la situazione anomala delle Regioni a Statuto speciale crea una situazione di iniquità difficilmente spiegabile ai cittadini delle altre Regioni e così assistiamo a fenomeni di vero disagio, che potrebbero addirittura sfociare in problemi di ordine pubblico nei territori di confine fra le Regioni a Statuto ordinario e quelle a Statuto speciale. Questa riforma riuscirà a produrre effetti benefici solo se metterà in piedi un sistema più chiaro, più semplice, più equo di quello attuale. Sul versante della riduzione degli sprechi sarà un'ottima arma nel momento in cui conterrà il principio secondo cui a una maggiore autonomia deve corrispondere una maggiore responsabilità. I due elementi dovranno essere inscindibili. Per responsabilizzare, promuovere il senso civico e, a cascata, ridurre l'evasione fiscale sarà tuttavia indispensabile - ribadiamolo - che il federalismo fiscale contenga norme chiare e semplici che permettano al cittadino di capire dove vanno a finire i propri soldi. Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione si muove nella direzione opposta. Non semplifica, ma complica. Già oggi, il sistema fiscale italiano è fra i più complessi del mondo e l'impressione è che, con le norme contenute in questo disegno di legge, la complicazione tenda ad acuirsi. Il contribuente, per capire dove andranno a finire i propri soldi, versati con tasse e tributi, dovrà districarsi in un insieme di meccanismi incomprensibili per i non addetti ai lavori. Quanto più logico e ovvio sarebbe stato prevedere un unico tributo proprio per ogni livello istituzionale, in modo semplice e chiaro! Ovviamente, il tutto compensato da diversi meccanismi di compartecipazione e perequazione dei maggiori tributi nazionali a favore delle autonomie territoriali, in sostituzione dei trasferimenti erariali. Per una questione di semplificazione e trasparenza sarebbe stato utile almeno togliere il complicato meccanismo delle doppie addizionali a favore dei Comuni, e anche non prevedere la novità delle aliquote riservate per le Regioni. Tutti quei meccanismi che impediscono al cittadino di comprendere dove realmente vanno a finire le tasse versate sono i veri nemici del federalismo perché rendono impossibile l'identificazione delle responsabilità! Faccio un esempio di semplificazione: i sindaci del Veneto stanno portando avanti una proposta semplicissima, che può essere attuata fin da subito, che chiede che ai Comuni venga riconosciuta, in sostituzione dei trasferimenti, una compartecipazione del 20 del gettito IRPEF prodotto dai rispettivi territori. La proposta del 20 per cento è modificabile, con una percentuale diversa, ma dobbiamo riconoscere che è un meccanismo semplice e di facile comprensione per il cittadino. Per quanto riguarda i Comuni, ritengo sciagurato quello che il Governo ha fatto sei mesi fa con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, senza che questa sia stata compensata con adeguati trasferimenti statali. Naturalmente tutto questo dovrebbe essere inquadrato nell'ambito di un Patto di stabilità intelligente, equo e razionale. Molto più razionale di quello attuale, che di fatto è uno strumento iniquo, bizantino e irrazionale. Proprio in questi giorni lo avete reso ancora più iniquo con le deroghe approvate a favore del Comune di Roma. Ho presentato alcuni emendamenti al testo al fine di prevedere un Patto di stabilità per gli enti locali equo e razionale. Mi auguro che le modifiche proposte vengano accolte. Concludo, signor Presidente. Oggi arriva in Aula questo disegno di legge che, in sostanza, in tema di federalismo fiscale, non è altro che una cornice che limita gli ambiti di intervento e mette i paletti per i futuri decreti attuativi. Non ci sono scelte coraggiose. Si accontentano tutti, anche quei territori che già oggi sono privilegiati. Nessun numero, nessuna aliquota. Tutto è demandato a successivi decreti che saranno firmati dal Ministro dell'economia, Ministro del quale peraltro non abbiamo potuto sentire il parere. Resta il timore che i decreti attuativi, se e quando arriveranno, non potranno stimolare quelle scelte che né il Governo, né il Parlamento sono stati in grado di fare fino ad oggi. Resta, fondatissimo, il timore che l'intero meccanismo possa inevitabilmente incepparsi. Inutile negarlo: questo testo porta con sé una serie di contraddizioni che non siete riusciti a risolvere perché in questi mesi siete stati occupati a tenere a bada le parti politiche della vostra coalizione contrarie alla riforma e lo avete fatto attraverso concessioni di tipo clientelare. Ricordo i 140 milioni di euro a favore di Catania, le deroghe al Patto di stabilità per il Comune di Roma, oltre al finanziamento eccezionale di 500 milioni di euro per lo stesso Comune. Se a questo aggiungiamo che avete voluto inserire nel testo del federalismo l'articolo che prevede l'istituzione di Roma capitale appare chiaro che questa riforma è frutto di una continua mediazione. Il federalismo può essere uno strumento per combattere le ingiustizie e le iniquità presenti nel nostro Paese, ma questo strumento può funzionare se viene costruito senza mediazioni irrazionali con effetti che moltiplicano le iniquità. Concludo Presidente, al nostro Paese serve un buon federalismo fiscale. Temo che il testo prodotto non riuscirà a darcelo. Temo che già dai primi decreti attuativi i veti incrociati e la indisponibilità a cedere quei privilegi che alcuni territori nel tempo hanno consolidato impediranno di fare le scelte necessarie all'interesse generale.

*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Ministri, ci troviamo ad affrontare oggi una seduta quasi storica. Non per enfatizzare il momento, ma oggi affrontiamo un disegno di legge che, nella sua formulazione e in tutta la fase di attuazione, uno sforzo forse non paragonabile ad altri fatti dal legislatore in questi sessanta anni di vita repubblicana. La stessa riforma tributaria degli anni 1971-1973, che fu una riforma sostanzialmente e fortemente modificativa dell'assetto preesistente, proprio con il suo obiettivo di centralizzare i tributi, pur istituendone di nuovi non ha determinato quegli scompensi e quelle difficoltà operative che indubbiamente sono insite in un processo così complesso, che dobbiamo però tendere ad eliminare in modo da renderlo efficace ed effettivo.

che il centrodestra ha sempre guardato con grande rispetto alla riforma del Titolo V, pur rappresentandosi da subito le difficoltà, le antinomie, le contraddizioni, la confusione che quella riforma avrebbe determinato, come poi è avvenuto. Già nel 2001 si è posto il problema di portare ad attuazione concreta quella riforma,

ancor più spedito e più semplice, considerando le ricadute che questo processo avrebbe determinato sulle istituzioni, sulle imprese, sulle famiglie, sui singoli cittadini. Quindi, si sposò il processo di attuazione e furono approvate leggi importanti: la legge La Loggia, ad esempio, che attuava parti significative della riforma del Titolo del Titolo V e che conteneva anche una norma di delega per riscrivere quel Testo unico degli enti locali proprio alla luce del nuovo modello che la Costituzione proponeva per gli enti locali. Fu approvata la legge Buttiglione che sostituiva la legge La Pergola, la cosiddetta legge che disciplina l'attuazione degli obblighi comunitari. Anche questo è stato un passo determinante perché si cercava di dare seguito alla riforma costituzionale rendendo adeguato il modello legislativo ordinario a quella riforma. Nel contempo, si mise mano anche ad una profonda riforma

dai cittadini, che però portava sul tappeto temi che anche oggi sono posti prepotentemente e sono iscritti nell'agenda politica: il problema, innanzitutto, di una semplificazione del quadro del federalismo. Infatti, chi ama e vuole perseguire questo nuovo modello di Stato e di rapporto tra cittadino e istituzioni sa benissimo dopo l'esperienza di questi anni che, se il rapporto è eccessivamente complicato e conflittuale, alla fine a prevalere è la ragione del più forte; non c'è più la ragione che impone la legge, ma la ragione del più forte che è lo Stato. pose inoltre il problema di creare il Senato federale, l'invocazione all'introduzione di una Camera federale nel nostro sistema, come si pose allora e si pone oggi fortemente e prepotentemente la necessità che, a fronte di un sistema aperto e forte di autonomie locali, ci sia un sistema di governo forte, responsabile, autorevole, ma non certamente autoritario. Quel tipo di riforma complessiva non passò, ma oggi alcuni di questi passaggi sono necessari, proprio per rendere meno complesso il percorso verso un federalismo compiuto. È necessaria quindi una una riscrittura, non tanto delle competenze regionali quanto dei rapporti e dei modi di attuazione di tali competenze, dei processi che portano

di intervento da parte delle leggi regionali che sono - e voglio un attimo replicare al collega che citava il mio intervento sulla questione pregiudiziale - l'altra faccia del federalismo. Infatti, il federalismo, anche quello fiscale, si pone soprattutto sul piano legislativo. I titolari delle funzioni legislative sono lo Stato, da una parte, e le Regioni, Le autonomie locali hanno importanti funzioni e prerogative, ma certamente non hanno la funzione legislativa.

normativo riammodernato, rivisitato e riequilibrato, quale potrebbe essere quello di un nuovo contesto normativo costituzionale. La Costituzione contiene inoltre delle ulteriori questioni che incidono sull'attuazione del federalismo: a parte il ragionamento sulle competenze confuse, ci sono le competenze variabili, quelle che aprono nuovi scenari. È necessaria quindi una normativa flessibile, ma anche una riflessione sull'articolo 116. Inoltre, abbiamo le autonomie speciali, le Regioni a Statuto speciale,

di un altro elemento che credo il disegno di legge abbia ben tenuto presente e che, in ogni caso, va ulteriormente approfondito in fase di attuazione. Non escludo che in un percorso di riforma costituzionale si possano individuare dei punti più fermi e più sicuri. Oltre il percorso costituzionale - e qui abbiamo avuto occasione di registrare anche da parte del Governo un impegno preciso, che credo si tradurrà a breve anche nell'approvazione di testi governativi - c'è il problema delle funzioni delle autonomie locali. Ho già accennato prima che una delle preoccupazioni che avemmo due legislature fa fu proprio quella delle nuove funzioni deiComuni, tant'è che la cosiddetta legge La Loggia conteneva una delega in questo campo. Tale delega non fu esercitata; forse era troppo ambiziosa, forse non era maturo ma comunque a questi temi occorre metter mano. Anche in questo caso occorre proporre un intervento che semplifichi e chiarisca il quadro sostanziale che deve essere tenuto presente dal legislatore fiscale nel momento in cui dovesse approvare i decreti legislativi. È un grande progetto. Ritengo sia senz'altro merito della Lega l'aver iscritto nell'agenda politica, con tempi precisi, il processo che oggi iniziamo iniziamo ufficialmente in quest'Aula. Credo anche che ogni spirito liberale non possa che condividere questa grande aspettativa, questo grande traguardo che è tipico di ogni Stato, dove si vuole mettere al centro del sistema pubblico il cittadino, in tal modo avvicinando e rendendo omologhi il centro di spesa ed il centro di entrata. Avvicinando i cittadini alle istituzioni

ampiamente condiviso e portare anche a un miglioramento del rapporto tra cittadini e istituzioni e anche tra cittadini e politica, perché maggiore trasparenza, consapevolezza possono essere elementi che aiutano ad avviare a soluzione la grande "questione morale" che colpisce in questo momento, ma non da oggi, le nostre istituzioni e la nostra attività politica.

L'attuazione del federalismo fiscale comporta il siglare un accordo in cui il concetto di solidarietà ne tessa le fila: il cittadino, in quest'ottica, mette a disposizione le proprie risorse nei confronti degli altri, in modo da far sì che il dovere verso lo Stato e verso la comunità più vicina consenta di determinare quella solidarietà orizzontale che affianca e rafforza la solidarietà verticale. In questi mesi, l'immanenza dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione si è trasformata in imminenza di risultato. All'interno della Commissione si è fatto molto anche il Partito Democratico ha contributo, a mio e nostro giudizio, in modo determinante. Crediamo, però, che si debba fare ancora molto. Ciò che serve è soprattutto un'armonia tra la riforma del federalismo fiscale, la Carta delle autonomie, l'attuazione degli articoli 114 e 117 della Costituzione e la riforma del Senato federale. Rischieremmo altrimenti, come è stato ben spiegato dal collega relatore Vitali, di dare nuovo carburante ad una macchina già vecchia, obsoleta e superata. In fondo, noi stiamo chiedendo molto ai cittadini, chiediamo soprattutto un atto di fiducia e dobbiamo essere in grado di dare gli strumenti e di consentire loro di capire dove vogliamo andare.

dell'Aula. Attraverso questa riforma, si tratta di riprendere anche un altro concetto, accanto ai tre principi cardine della individualità, della progressività e della centralità: si tratta di coniugare, sostanzialmente, l'articolo 53 della Costituzione con l'articolo 29 della stessa, quindi cercare anche di porre in essere la capacità contributiva individuale insieme a quella della comunità familiare. Questo è un altro punto aperto sul quale il Partito Democratico ha dato un contributo non indifferente grazie all'introduzione nel testo iniziale del patto di convergenza, attraverso il quale il passaggio dalla spesa storica ai costi standard per le Regioni dà la possibilità alle stesse di offrire ai cittadini maggiori servizi, quali gli asili nido o alcuni servizi di carattere scolastico. Dobbiamo cercare di sanare quello squilibrio territoriale nell'offerta dei servizi così da coniugare meglio quelle tre parti dell'Italia. Noi crediamo, comunque, che il federalismo sia ormai una scelta matura, capace di coinvolgere tutti, dai singoli cittadini, agli enti territoriali, alle istituzioni centrali. Proprio in questa *liaison*, per alcuni forzosa e per altri cercata e voluta, sta anche la grandezza di questo provvedimento. Certo, resta un *punctum* *dolens* all'interno di questo dibattito e credo che anche alcuni esponenti della maggioranza riconoscano questa nostra osservazione. La prima scelta del Governo, quella di abolire l'ICI, che pesa per circa il 25 per cento sul gettito complessivo, non è andata sicuramente in questa ha tolto l'unica imposta locale. Sarebbe quindi doveroso che in questa sede il Governo mettesse a disposizione le risorse compensative adeguate per offrire le risorse necessarie agli enti territoriali ad affrontare i cambiamenti. Occorre anche - e per noi del Partito Democratico è indispensabile - che l'ambito dell'autonomia tributaria degli enti territoriali sia ben definitiva, perché non si può essere approssimativi su questo tema, ma occorre un *numerus clausus* che non lasci spazio ad interpretazioni. Fino ad oggi, l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione ha confermato la sperequazione tra le Regioni del Nord e del Sud, non ha uniformato e corretto la diversa qualità e quantità dei servizi al cittadino e soprattutto ha accentuato la diffidenza del cittadino nei confronti dell'amministrazione delle risorse pubbliche. La vera sfida, quindi, è quella di permettere ai cittadini di avere gli stessi diritti dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, senza doversi spostare per ottenere, il vero termine di confronto. La famiglia e il cittadino devono restare il fulcro del provvedimento, a cui poter assicurare livelli essenziali di prestazioni civili e sociali, occorre stabilire quali siano e poi lasciare alle Regioni la scelta di plasmarli a seconda delle necessità locali. Appare quantomeno discutibile che il Governo abbia deciso di escludere il trasporto pubblico e che non sia chiaro se l'edilizia scolastica rientri oppure no nei livelli essenziali di prestazione. Sarebbe bene, dunque, se anche grazie a questo dibattito, che mi sembra pacato e sereno, si chiarisca tale punto.

che ci permetterà di controllare i decreti attuativi, purché attraverso il suo Regolamento interno essa sia indipendente: sul punto vogliamo essere molto chiari!

i modi più opportuni ed adeguati per l'edificazione e lo sviluppo di una società adulta e solidale, attraverso una più efficace articolazione della convivenza, che faccia crescere la qualità

sappiamo che nell'opinione pubblica con il termine federalismo si intendono tante questioni. Esso viene considerato come uno strumento per porre rimedio a deficit strutturali del nostro Paese. Vi è il tema della questione fiscale, uno scambio ineguale che in molti territori viene avvertito tra ciò che il cittadino dà alle istituzioni pubbliche e ciò che riceve in cambio. Vi è poi il grande tema della pressione burocratica, che a volte pesa per la vita delle aziende più di quanto possa contare la pressione fiscale. Vi è il tema di una inefficiente perequazione: quella solidarietà tra territori che non produce risultati apprezzabili di ammodernamento e di elevamento della prestazione dei servizi. Vi è l'evidente distorsione del sistema di trasferimento

Calabria 490 euro e uno della Sicilia 570 euro, ci rendiamo conto che c'è una sperequazione inaccettabile tra i cittadini. Ritengo che vi siano molte aspettative sulla prospettiva di passare ad un sistema in cui il federalismo diventi uno strumento di soluzione e penso perciò che un fallimento fallimento trascinerebbe con sé non solo la maggioranza, ma tutta la credibilità delle istituzioni. Per tale ragione ci siamo impegnati a suo tempo con l'approvazione del Titolo V e ci siamo impegnati in questo passaggio per proporre le modifiche che ritenevamo necessarie. Credo che ci siano due grandi questioni politiche da affrontare.

un differenziale così elevato. Attenzione: non è il livello di governo che giustifica questo differenziale. Ci sono servizi interamente gestiti dallo Stato (è il caso della scuola)

Oppure ci sono servizi interamente affidati alla responsabilità decentrata delle Regioni (pensiamo alla sanità), in cui pure permangono fortissimi differenziali di efficienza. La seconda grande questione occorre un nuovo patto nazionale di redistribuzione delle risorse. Quello che c'è non regge più. Semplificando un po', diciamo che non regge al Nord. non regge al Nord. È vero che il Nord è la parte più ricca del Paese, ma è anche la parte che deve affrontare le più intense trasformazioni. Il sistema delle autonomie locali è sotto stress perché c'è un forte innalzamento dei livelli di richiesta di nuovo *welfare*. Penso al forte invecchiamento delle popolazioni alla forte trasformazione della base sociale delle comunità locali, con nuovi cittadini che entrano nel territorio nazionale. Ricordo, solo a titolo di esempio, che nel mio territorio ci sono dati sull'affluenza scolastica che dimostrano che, in molte scuole elementari, il 40 per cento degli iscritti sono bambini nati fuori dal territorio italiano o nati in Italia da genitori stranieri. inoltre al grande tema della qualità delle nostre città e al loro degrado. C'è quindi una nuova richiesta di servizi e, insieme, lo stress di molti territori, alle prese con una fortissima competitività internazionale che richiede nuove infrastrutturazioni. Ma questo patto non regge neanche al Sud. Il*surplus* di trasferimenti realizzato con queste regole non ha prodotto, per quei cittadini e per quei territori, nuovi servizi e nuove capacità competitive.

po' no. Voglio anch'io dare atto ai ministri Bossi e Calderoli di aver fatto una scelta saggia e di aver compreso non solo che, in materia di regole e di quadro costituzionale, è bene che si trovi un'intesa, ma anche che, poiché il percorso del federalismo sarà lungo e richiederà il consenso di una pluralità di istituzioni, tanto più può essere solido questo percorso quanto più solide e condivise sono le sue fondamenta. In questo caso la scelta del Governo è stata netta e noi ne diamo atto volentieri. Penso che se questa

piuttosto assenti nel sistema istituzionale italiano. Il sistema dei costi standard con il patto di convergenza, che abbiamo proposto e che è stato introdotto, indubbiamente adempie a questo obiettivo e nel tempo sarà capace di produrre dei risultati importanti. Tuttavia, anch'io devo

non credo ci sarà l'adeguata semplificazione e trasparenza fiscale che rappresenta uno degli elementi importanti di un sistema federale. Resta, purtroppo, un sistema molto barocco,

la complessità che, purtroppo, resta. Poi, naturalmente, manca la parte istituzionale. Anch'io sono convinto che senza la Carta delle autonomie che ridefinisca il sistema dei poteri locali, le competenze e il Senato federale,

si tiene nella misura in cui, in attesa del federalismo che verrà e che richiede tempi lunghi, troppo lunghi rispetto a quanto io penserei necessario per il Paese,

tra il federalismo promesso e proclamato e le scelte di tutti i giorni, che vanno in direzione di una diminuzione degli spazi di autonomia

se sarà un federalismo municipale. Le politiche fin qui adottate in direzione di una compressione dell'autonomia e della capacità di azione dei Comuni

di non dover più vedere attuate, nel frattempo, politiche distruttive dell'autonomia dei Comuni e di quei principi di merito, di responsabilità che sono la base di un moderno municipalismo.

il federalismo fiscale apparentemente è un concetto abbastanza semplice: della discussione pubblica e della discussione parlamentare. Si è infatti partiti da un inizio forse un po' farraginoso in cui appariva come la proiezione di un modello che è stato detto - forse erroneamente - lombardo, al quale il federalismo si qualificava come una sorta di realizzazione di un meccanismo per cui le Regioni si tengono le proprie risorse,

ha assunto la forma di un progetto di semplificazione dell'armatura fiscale dello Stato. Se dovessi spiegare a degli studenti che cos'è il federalismo fiscale, comincerei dicendo che è il tentativo di

non c'è nessun orgoglio di parte nel rivendicarlo: quella riforma è stata bocciata sì da una maggioranza di centrosinistra, ma con il contributo fondamentale e prezioso - e che bisogna riconoscere in pieno - di una parte significativa dell'elettorato di centrodestra, che non si è riconosciuta in quel disegno e che ha preferito salvaguardare la Costituzione com'era, piuttosto che ritrovarsi una Carta costituzionale dubbia, così com'era stata progettata.

con un spirito differente, più dialogico e più interlocutorio, una proposta di federalismo fiscale e non una riforma generale della forma dello Stato.

C'è chi ha pensato che per realizzare il federalismo fiscale si dovesse prima cambiare di nuovo tutta la configurazione di Regioni, enti locali, rapporti con lo Stato e così invece, abbastanza positivo il fatto che stiamo dibattendo del federalismo fiscale senza dover oggi - e spero anche domani e domani l'altro - discutere di una nuova riforma globale della configurazione dello Stato. Stato. Ognuno ha le sue ragioni da affermare ed io voglio dire la mia, perché ritengo che ciascuno debba esprimere anche dei punti di vista all'interno del proprio schieramento, con qualche tono particolare.

anche perché l'esperienza attuale ci dimostra che non c'è nessun bisogno di rafforzare il potere esecutivo: è già abbastanza forte, troppo forte, e quello specifico di oggi è rafforzato da un potere extraistituzionale che in nessun'altra democrazia sarebbe accettato. È meglio quindi fermarsi qui.

dovremo impegnarci per fare in modo che non si determini una complicazione del fisco. Vi è poi la questione della sperequazione tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario: anche questo è un aspetto che pesa sull'orizzonte della discussione.

la ricchezza di una Nazione è costituita anche da moltissimi e diversi elementi che, pur non essendo tutti direttamente monetizzabili, non per questo hanno minor rilievo. C'è una parte della ricchezza della Nazione che è difficilissimo tradurre in euro,

che gestisce la captazione del vento - che è di tutti - e che dà alla Regione e ai locali le briciole delle briciole. di questo tipo non rientra nel calcolo del federalismo fiscale, ma essendo quest'ultimo un processo di semplificazione dell'uso delle risorse, non può alla lunga non tener conto di queste formidabili e insidiose diseguaglianze che si attestano nella gestione del territorio. quindi che, andando avanti in questo processo di semplificazione, il nostro compito d'iniziativa propositiva e positiva è quello di tener che bisogna salvaguardare i beni comuni: non sto ad elencarli perché li avete tutti ben presenti di fronte a voi. La speranza e il pessimismo si possono combattere in una forma incerta: si può essere ottimisti, si può essere pessimisti. Io penso che oggi che ci siamo impegnati in quest'opera di contribuzione propositiva a modificare la legge dobbiamo avere un atteggiamento positivo, quindi non possiamo permetterci un eccesso di pessimismo; però devo osservare che la prassi di Governo non incoraggia questo tipo di orientamento positivo, perché le cose perché le cose avvenute sotto i nostri occhi testimoniano una dilapidazione spaventosa di risorse che potevano essere utilizzate in maniera molto più significativa

essere utilizzati in altro modo. In ultimo, l'Italia dei Valori si propone, in base a questo atteggiamento propositivo e positivo, di svolgere essenzialmente proposta e sorveglianza democratica. La sorveglianza democratica deve essere rivolta al al vuoto virtuale creato dai decreti delegati. Questa è una legge delega, di cui molti hanno detto che è una scatola chiusa: io non penso che sia così, però potrebbe rischiare di esserlo. Se la legge delega sarà risolta da decreti delegati su cui il Governo eserciterà un dominio totale, senza il controllo e la possibilità d'interlocuzione dell'opposizione, l'Italia dei Valori, insieme al Partito Democratico,

un disegno di legge che, se può essere ampiamente condiviso nelle finalità, ha presentato degli elementi di criticità, tant'è che, fra la prima e l'ultima stesura, frutto di un paziente lavoro degli ottimi ministri Calderoli e Bossi, del relatore e delle Commissioni, vi sono differenze notevoli con correzioni tecnico-giuridico di non poco conto, a partire dall'articolo 5 che nei contenuti era stato abbondantemente superato dall'abrogazione contenuta nelle leggi Bassanini, nel Titolo V novellato e nella legge cosiddetta tutte discipline che hanno stabilito che il decentramento territoriale italiano si fonda sul finanziamento delle funzioni pubbliche e non su quello delle materie appartenenti a Stato e Regioni e soprattutto hanno prescritto che la competenza amministrativa generale inerente l'esercizio di tali funzioni spetta ai Comuni e non alle Regioni. Un rilievo di principio va fatto sulla non comprensione che il sistema costituzionale attuale non è un federalismo classico, ma una sorta di municipalismo spinto. Finalmente, il testo emendato alla nostra attenzione ha colto un aspetto fondamentale del Titolo V: V: l'attuazione dell'articolo 119 non è effettivamente e concretamente realizzabile se non si definiscono le funzioni fondamentali dei Comuni secondo quanto stabilito dall'articolo 117. Ciò che forse non si comprende è che, nonostante la riforma si intitoli enfaticamente: «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale», il sistema costituzionale italiano riformato dal Titolo V non è un sistema federale classico, ma uno «Stato regionale a tendenza municipale», ovvero una «Repubblica delle autonomie». La Costituzione ha infatti posto sullo stesso piano Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e ha conferito un particolare rilievo proprio all'ente Comune, stabilendo che «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni», con la possibilità di attribuire le funzioni agli enti superiori solo nel rispetto del principio di sussidiarietà. C'è stata - starei per dire - una sorta di «calo di attenzione» dei redattori del testo nei riguardi dell'ente Comune, anche se questa oscurità sembra essersi diradata regolando l'ordinamento di Roma Capitale. Non solo si sono elargite gratuitamente significative porzioni di patrimonio statale alla città di Roma, ma le si sono conferite una serie di funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 118, tra le quali vorrei menzionare la protezione civile, la difesa dall'inquinamento, lo sviluppo economico-sociale, ossia funzioni che andrebbero definite come fondamentali e non certamente amministrative. Quando il legislatore costituzionale ha previsto l'ordinamento speciale di Roma capitale, non aveva di certo in mente di attribuire alla sola Capitale le prerogative che abbiamo ricordato, ma aveva posto i Comuni tutti Sarebbe stato semplicemente opportuno ritornare alla legge La Loggia e ricordare la funzione fondamentale del Comune e il principio di sussidiarietà verticale. Invece registriamo aggiunte posticce al disegno, peraltro in modo provvisorio, generando di conseguenza una serie di evidenti sfasature, senza contare che la regolamentazione di Roma capitale contenuta nel disegno genera una vera e propria disuguaglianza fra la città di Roma e gli altri Comuni capoluogo ed anticipa inopinatamente, di fatto, quel federalismo istituzionale che sarebbe dovuto partire in parallelo con il federalismo fiscale per rendere credibile ed efficace la riforma. la riforma. L'articolo 2 del nuovo testo introduce il superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di un costo e fabbisogno standard cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni; un obiettivo altamente condivisibile, volto a ridurre gli sprechi e le spese gonfiate. Vorrei sottolineare che il Sud deve considerare tale obiettivo come una opportunità di sviluppo e non certamente come una *deminutio*. Spetta infatti a noi meridionali selezionare finalmente una classe dirigente capace e politicamente responsabile nell'utilizzo delle risorse derivanti dalla tassazione; una classe dirigente capace di attrarre le risorse europee senza lasciarle agli altri Paesi; una classe politica in grado di creare opportunità per accrescere le ricchezze locali; una classe dirigente che non chieda soltanto danaro ma che sappia innanzitutto dimostrare di saperlo utilmente impiegare. Ogni amministratore politicamente responsabile del Sud Italia, in altre parole, dovrebbe avere come principale obiettivo quello di ridurre progressivamente, sino ad eliminare, le somme erogate dal fondo perequativo. Su questo credo siamo tutti d'accordo; peccato che non sia così semplice e soprattutto immediato nel nostro Meridione, vuoi per carenza di classe dirigente, vuoi per evidenti disparità infrastrutturali, vuoi per l'irrisolto problema della criminalità che scontiamo a causa di uno Stato per troppo tempo assente e disattento. Tutto ciò accade pur in presenza di qualche capace amministratore del Sud che non può operare nelle condizioni migliori. Veniamo per un attimo al principio della territorialità. Abbiamo sottolineato più volte come sia cruciale che il calcolo sulla compartecipazione ai tributi erariali sia effettuato tenendo conto del luogo dell'effettivo consumo o dell'esecuzione della prestazione e non unicamente di quello della residenza fiscale. Se così non fosse, vi sarebbero innumerevoli esempi di sperequazioni fra Nord e Sud, nel senso che la tassazione del contribuente del Nord che svolge la propria prestazione al Sud non verrebbe calcolata come ricchezza del Sud, in quanto dichiarata nel suo luogo di residenza. Il nuovo articolo 7, riformato dalle Commissioni riunite, introduce in effetti il luogo di consumo per i tributi aventi quale presupposto i consumi, precisando che per i servizi il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale. Il limite di tale previsione è che essa è stata introdotta soltanto in ordine alle modalità di attribuzione delle compartecipazioni ai tributi erariali delle Regioni e non anche dei Comuni, ancora una volta dimenticando che le funzioni fondamentali e amministrative spettano per definizione ai Comuni e non alle Regioni, come prevede il nostro sistema costituzionale. Ciò premesso, ho ritenuto per l'appunto di proporre la medesima norma anche a favore dei Comuni presentando un emendamento, in modo da ricomprendere tutte le ipotesi in cui il territorio del Sud è utilizzato dalle imprese del Nord soltanto - lo dico chiaramente - a fini di sfruttamento (gli esempi sono innumerevoli: potrei citare l'ILVA di Taranto, le società che gestiscono parchi eolici e tante altre situazioni che esistono nel nostro Sud). Un'altra incomprensibile *deminutio* per il Sud deriva, a mio parere, dalla mancata previsione della funzione di cassa a livello dei territori. All'articolo 2 si prevede che i tributi erariali compartecipati siano integralmente contabilizzati sul bilancio dello Stato. L'articolo 119 della Costituzione prevede che le funzioni pubbliche siano finanziate, fra l'altro, dalle compartecipazioni ai tributi erariali versati sul territorio, ossia trattenendo le relative risorse sul territorio ove vengono versate, così da finanziare direttamente ed immediatamente le funzioni pubbliche comunali. Ma il testo in discussione è ancora ondivago. Da un lato, è stato richiesto a tutti livelli di governo di essere istituzionalmente leali gli uni con gli altri, affinché tutte le amministrazioni pubbliche concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai Trattati internazionali, ma, dall'altro, si è mantenuta l'unicità contabile del "Centro", prevedendo che i tributi erariali compartecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato. La lealtà richiesta comporta che Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni adottino per le proprie politiche di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità e crescita, sicché gli enti debbono essere messi nelle migliori condizioni di poter rispettare i rigidi vincoli imposti dal Patto di stabilità. Facciamo l'esempio dell'IRPEF: su una base ipotetica di 100 di IRPEF, della quale 60 deve essere assegnata agli enti locali, nel bilancio dello Stato verrà iscritta una voce di entrata pari a 100, salvo poi indicare il trasferimento di 60; di contro, nel bilancio degli enti locali avremmo un'entrata pari a zero e un trasferimento per 60. È abbastanza evidente che così procedendo diviene arduo rispettare i vincoli di saldo fra entrate e spese previsti dal Patto, mentre sarebbe più corretta una contabilizzazione di ciascuna quota da parte degli enti di competenza, 40 nel bilancio dello Stato, 60 nel bilancio degli enti. I principi di conoscenza e di unitarietà delle poste iscritte in bilancio possono invece essere assicurati dall'apposita previsione di un allegato al bilancio dello Stato dove vengono riportate integralmente le somme derivanti dai tributi erariali compartecipati. È questo il senso che si evince dall'articolo 119 della Costituzione. Tutto ciò scoraggerebbe i sindaci dall'essere virtuosi, perché da un lato si introduce il costo standard delle prestazioni, dall'altro non si consente agli enti territoriali di usufruire in tempo reale delle somme derivanti dalla compartecipazione e gli inevitabili ritardi nella procedura di ritrasferimento si ripercuoteranno negativamente soprattutto sul Sud Italia, notoriamente zona più povera. Infine, non poche perplessità desta la cosiddetta perequazione infrastrutturale, che rischia di produrre i suoi effetti fra anni, dopo che, attraverso le delibere CIPE, i fondi per le aree meno dotate di infrastrutture saranno stati dirottati altrove. In conclusione, il provvedimento è importante, condivisibile in linea di principio, un'opportunità per il Meridione, ma se resta così com'è rischia di essere condizionato dalla mancata attuazione della parte istituzionale del Titolo V e dalla mancata realizzazione del principio di sussidiarietà. Ci auguriamo che in un lavoro comune, nella continuità delle norme dalla Bassanini alla legge La Loggia, anche l'Aula possa fare la sua parte per esitare un testo che sia più condivisibile e più adeguato alle finalità volute e che configuri una vera uguale linea di partenza per una leale competizione fra territori, nella quale avrà la meglio chi saprà interpretare più attivamente le istanze identitarie territoriali con onestà, lucidità programmatoria ed alto senso di responsabilità.

casuale - sulle vicende relative alla questione di Roma capitale. Lo faccio per un'idea opposta a quella di chi adesso mi ha preceduto. È vero, vi è necessità di dare alla capitale del Paese una sua configurazione più precisa; è un argomento sul quale il dibattito va avanti da anni: alcune condizioni la Costituzione le ha progressivamente create, ora bisogna agire.

definito, che tra l'altro mettesse insieme la vicenda delle aree metropolitane, la questione di Roma capitale, lo sviluppo armonico di un'area come quella romana all'interno di una comunità più vasta, che è quella nazionale, ma che è anche quella della Regione Lazio in particolare. Si è scelta invece una strada diversa: quella di introdurre un emendamento, preparato nottetempo nell'approvazione del disegno di legge a Palazzo Chigi, che poi ha subito una serie di ritocchi. Il risultato di questa fretta si vede: siamo di fronte ad un provvedimento indefinito, appunto per quanto riguarda le ragioni della capitale, e frettoloso. Chi come me ama questa città - ho avuto l'onore ed il privilegio di servirla come amministratore per tanti anni - non può che provare amarezza e allarme per una vicenda che vede in atto nei fatti uno scambio politico tra alcune ragioni del federalismo e gli interessi di chi questo federalismo non vuole votare e magari nella maggioranza si fa scudo di qualche potere in più per Roma capitale e per il sindaco della città. Ci si ricorda costantemente che Roma è la più grande area comunale d'Europa, che è una città estesissima (lo sappiamo bene tutti); ci si ricorda che nella stessa ogni mattina circolano 4 milioni di persone, di cui quasi uno viene da fuori per ragioni di pendolarismo, si rinunzia, a fronte di una situazione come questa, a governare questa entità così grande con un governo di area più vasta. appunto, la via subordinata, transitoria (e lo sappiamo nel nostro Paese come vanno le questioni transitorie), destinata a durare un tempo indefinito, come indefinita è la normativa che esce dal dibattito nella maggioranza e dal lavoro delle Commissioni. Noi volevamo non un provvedimento così debole ed indefinito. Volevamo che si discutesse per Roma capitale di uno sviluppo organico della città con i territori e le comunità circostanti, quali quelle della Provincia di Roma, dei paesi che - voglio ricordarlo - insistono su quest'area da prima della nascita della città di Roma, dell'intera comunità regionale.

si fa un elenco numerico di alcuni elementi (su ciò richiamo ancora l'attenzione del Governo e di noi legislatori perché non si costruisca una cosa che non sta in piedi) è la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali. Domando allora a tanti di noi che hanno fatto gli amministratori: quando in genere parliamo nell'amministrazione comunale di valorizzazione, parliamo di qualche cambio di destinazione d'uso per la vendita, per la messa a reddito; qui parliamo del patrimonio artistico più importante del mondo, come spesso ci ricordiamo nelle premesse di queste leggi e nelle relazioni o nelle lettere che il nostro collega vice sindaco di Roma ci manda in occasione degli auguri di Natale; e allora, che facciamo? Come lo valorizziamo? Cosa intendete per "valorizzazione"? Perché non allegate una chiara relazione? Ripeto: Roma ha bisogno di interventi di conservazione importanti, della tutela dello Stato; chiariamo che cosa vuol dire "valorizzazione", perché c'è il sospetto che sia il tentativo di fare senza controlli magari qualche corsa delle bighe da qualche parte. E pensiamo al rischio che, invece di aver fatto una legge per Roma capitale, avete cercato un compromesso al ribasso che o è inutile, perché è già contenuto nelle leggi esistenti (vedi il turismo, eccetera), o rischia di essere un colossale imbroglio perché sotto banco inserisce qualcosa che non capiamo. Lo stesso discorso vale per il punto *b)* del medesimo articolo, nel quale introducete il tema della VIA: cioè, al Comune di Roma viene attribuita la valutazione di impatto ambientale.

sappiamo come va a finire nel nostro Paese quando si allenta il sistema dei controlli su materie tanto delicate. Si dà tanta enfasi a Roma capitale, all'idea che bisogna compiere per questa città scelte complicate,

Se così la presentate e se così la volete approvare, è chiaro che non c'è la nostra disponibilità a votarla, come cittadini di questa città, come amministratori e come legislatori responsabili; di affermare che avete fatto un pasticcio sotto il quale rischia di nascondersi qualcosa di molto grave. Signor Presidente, se è vero che le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica (come prevede l'articolo 119 della Costituzione), è anche vero che da troppo tempo è mancata l'attuazione legislativa di questa norma costituzionale. Il federalismo fiscale oggi al nostro esame conferisce finalmente certezza normativa a tutte le Regioni del Nord, come a quelle come a quelle del Sud. Nel dibattito pubblico e nella pubblicistica ormai consolidata su questo tema c'è stata fino ad oggi una contrapposizione territoriale tra chi ha rivendicato il ruolo delle Regioni del Nord e chi invece, in nome di un meridionalismo storicamente superato, ha lamentato le presenti carenze dello Stato verso le Regioni del Sud: cioè, alla "gramsciana" questione meridionale è stata di recente contrapposta la questione settentrionale. Il dibattito è andato avanti per anni, fino ad oggi, dividendo l'opinione pubblica in una contrapposizione netta che è diventata quasi tra due tifoserie, una per il Nord e l'altra per il Sud. oggi in quest'Aula viene superata, grazie ad un'intesa politica che è intervenuta nella coalizione di centrodestra tra il Popolo della Libertà e la Lega, e si è potuti giungere ad un disegno di legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Occorre dire che con questo disegno di legge del Governo si attua direttamente il dettato costituzionale, si dà rilievo a interventi a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, ma - e qui è la novità sostanziale - li si disciplina con una legge, con la conseguenza, quindi, di introdurre anche un maggiore controllo sui trasferimenti alle Regioni più svantaggiate. In altri termini, sono giuste la solidarietà e la coesione sociale (come scritto nell'articolo 1 del testo), ma che siano finalizzate a creare uno sviluppo vero per le aree svantaggiate del Paese: solidarietà utile e non più assistenzialismo fine a se stesso. Ma quel che vorrei sottolineare è anche quel "mix" di diritti e doveri che - con il federalismo fiscale - le singole Regioni assumono di fronte ai propri elettori- contribuenti. Il disegno di legge va considerato un'opportunità di crescita economica ma anche un'occasione di recupero e consolidamento dei vincoli di trasparenza e di correttezza amministrativa tra cittadini e Regioni. Allora, l'obiettivo è di assicurare autonomia di entrata e spesa agli enti locali e di sostituire il criterio della spesa storica con quello dei costi standard. L'obiettivo è quello di arrivare a una complessa diminuzione della pressione fiscale, prevedendo che sia garantita, attraverso i decreti attuativi, la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale, nonché del suo riparto tra i vari livelli di governo. Ancora, viene introdotta la previsione del coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione fiscale. Sono previste sanzioni fino al commissariamento per Comuni, Province e Regioni inadempienti e un sistema premiale per gli enti virtuosi. locali fanno ricorso per l'erogazione dei servizi al fondo perequativo, alla compartecipazione ai tributi erariali e ai tributi propri, tutto quello che nel corso degli interventi che mi hanno preceduto è stato già indicato e delineato, anche se da punti di vista a volte contrapposti. Un altro punto di novità è quello del patto di convergenza: il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, individua un percorso dinamico di convergenza ai costi e fabbisogni standard, detto appunto "patto di convergenza", presentato insieme al Documento di programmazione economica e finanziaria alle Camere e che gli enti sono tenuti a rispettare. Trattandosi di una legge delega al Governo assumerà un valore essenziale la fase attuativa dei decreti delegati. Ecco allora l'istituzione di una Commissione bicamerale, così come indicato anche qualche mese fa dal presidente della Camera Fini, composta da senatori e deputati indicati dai Gruppi e nominati dai Presidenti delle Camere. Indubbiamente, un sistema federale è più vicino alle necessità delle persone e

una volta stabilito il criterio territoriale del rapporto tra amministrazioni locali e cittadini elettori-contribuenti, non devono essere perdute di vista questa situazione e le macroscopiche differenze che ancora oggi si verificano su questo argomento. Sarà allora opportuno contemplare la previsione di facilitazioni fiscali per le donne che lavorano con una connessione vincolante alla realtà locale. per questo motivo il federalismo fiscale deve rappresentare, proprio per l'importanza che rappresenta, un'opportunità da cogliere anche per riaffermare e promuovere l'occupazione femminile. Esistono realtà diversissime. I livelli più elevati di occupazione femminile e i più bassi differenziali tra uomini e donne si osservano nel Nord del Paese, in particolare in Emilia-Romagna dove il tasso di occupazione femminile è pari al 60 per cento. Nel Mezzogiorno, i livelli sono molto inferiori e i differenziali differenziali di genere molto elevati. In Puglia, il tasso di occupazione femminile è meno della metà di quello dell'Emilia Romagna ed è due-tre volte più basso di quello maschile. È di tutta evidenza che di di questo noi dobbiamo tenere conto. Io ho presentato, con la senatrice Adamo, una serie di emendamenti in Commissione e devo ringraziare il Governo,

17, recante coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livello di Governo, che prevede, al comma 9, un sistema premiante per gli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità Mi auguro anche che, in sede di approvazione definitiva da parte dell'Aula del disegno di legge, si possa inserire in modo esplicito, approvando un emendamento che ho ripresentato per l'Aula, un riferimento al principio di pari opportunità, proprio in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione. Quando il Parlamento è in procinto di varare una riforma così importante come quella relativa al federalismo fiscale, è indispensabile che venga ricercata la più larga convergenza tra maggioranza ed opposizione. Nell'avviare il federalismo, ovvero nella determinazione dell'autonomia tributaria delle singole Regioni, si deve assolutamente evitare, quando si darà corso alla riforma, che si possano acuire le distanze

più evidente il rapporto tra prelievo tributario e servizi forniti e ciò non potrà che influenzare positivamente le entrate tributarie, con la conseguenza che sarà più difficile occultare completamente all'organo accertatore la fonte produttiva del reddito, data la descritta vicinanza tra controllore e controllato. È quindi fondamentale realizzare un maggior coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle procedure di accertamento. Dovranno entrambi smettere di vivere dei trasferimenti erariali, avendo solo capacità di spesa. Dovranno piuttosto cominciare a preoccuparsi del recupero delle imposte utili a finanziare i servizi da loro forniti a livello decentrato. A questo scopo è necessario potenziare l'anagrafe tributaria, intesa come l'insieme di tutti i rapporti tra Erario e contribuenti, che possono essere tracciati in maniera agevole grazie allo strumento telematico. Occorre fare in modo che le diverse banche dati,

che introduce un articolo che amplia le competenze della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, estendendone il controllo sulla gestione dei servizi di accertamento e sulla riscossione dei tributi locali. locali. Il federalismo, quindi, non significa e non deve significare spaccatura del Paese e contrapposizione netta tra Regioni avanzate e Regioni meno progredite; non significa divisione e conflittualità, ma gestione più equilibrata delle risorse, per avere più denaro a disposizione per fare funzionare meglio i servizi da rendere ai cittadini. Al

la prego di concludere. del Parlamento che il presidente della Camera Gianfranco Fini ha già indicato come via d'uscita per una migliore collaborazione tra maggioranza e opposizione, quella centralità del Parlamento che unisce i cittadini, che sono anche contribuenti, e non divide il Paese secondo calcoli di contrapposizione il passaggio che si sta compiendo è sicuramente rilevante. Si pongono le basi di un vasto, impegnativo ed estremamente complesso riordino del sistema di finanza pubblica da cui ci si attendono conseguenze importanti ed innovative. Il federalismo fiscale, come noi lo concepiamo, è una grande opportunità per modernizzare il Paese, riformare l'amministrazione pubblica, promuovere lo sviluppo dei territori. È anche una modalità utile a favorire la partecipazione dei cittadini al controllo della cosa pubblica per rafforzarne il rapporto fiduciario con le istituzioni e conseguire, attraverso il nesso di maggiore autonomia e più marcata responsabilizzazione degli amministratori a tutti i livelli di governo, maggiore economicità ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili. Introduce fattori positivi e temperati di concorrenza innovativa tra le diverse comunità e i governi locali, senza per questo abdicare al principio per cui il sistema pubblico nel suo complesso deve essere in grado di garantire l'esercizio dei diritti sociali e civili su tutto il territorio nazionale. Il federalismo fiscale non deve dunque diventare un tema di scontro da usare per ridurre il grado di coesione della collettività nazionale, ma anzi deve essere il perno attorno a cui saldare autonomia e solidarietà, un collante che aiuti a ricomporre, nella gradualità del processo della sua attuazione, i divari Nord-Sud quanto a dotazione di infrastrutture e servizi, oltre che ad amalgamare maggiormente le dotazioni dei territori all'interno delle diverse Regioni.

e, come ha detto il senatore Morando, è abissalmente lontano dal testo proposto dalla coalizione di centrodestra nel programma della sua campagna elettorale. Si è sviluppato un buon livello di confronto parlamentare, c'è stata apertura al dialogo e disponibilità a recepire contributi e rilievi critici dell'opposizione. Il risultato è un testo della delega meno ambiguo nei principi e più strutturato nel percorso di adozione dei decreti legislativi e per l'entrata a regime. Soprattutto, si è superato il pericolo di una rappresentazione statica, non dinamica ed evolutiva, del processo che deve superare la spesa storica per attuare un sistema di erogazione di servizi e funzioni a costi standard, per fabbisogni ed obiettivi standard; lo strumento del patto di convergenza, frutto delle nostre proposte innovative, ne costituisce il meccanismo insieme regolatore e propulsivo. Tuttavia, se il lavoro parlamentare è stato positivo (a dimostrazione che senza atteggiamenti di arroganza e chiusura pregiudiziale il confronto con l'opposizione è non solo possibile, ma utile, anche perché da parte nostra sono venute risposte costruttive e di merito), molti elementi sono ancora troppo vaghi e c'è l'alea di una traduzione delle intenzioni e del modello con esiti dai contorni molto incerti e problematici. pesato e pesa, nella discussione, la mancanza di un adeguato quadro di dati statistici attendibili, indispensabili per permettere una valutazione quantitativa e, soprattutto, qualitativa della posta in gioco. Come si verrà a scomporre nelle sue varie parti il gettito dei tributi? Quali dimensioni dovrà raggiungere il finanziamento perequativo? In rapporto a quale ottimizzazione dei livelli delle prestazioni e su quali tipologie di funzioni verranno parametrate le risorse disponibili? Tutto questo non ha risposte al momento. Considero un risultato della nostra tenacia nel sottolineare queste lacune il fatto che nel testo sia stato introdotto il principio di una relazione tecnica e finanziaria da accompagnare al primo decreto legislativo (previsto entro dodici mesi dall'approvazione della legge delega), per poter dare trasparenza al Parlamento, agli enti coinvolti e all'opinione pubblica circa le implicazioni e le ricadute di carattere finanziario e fiscale che conseguiranno dall'attuazione delle nuove norme. Non è molto, certo. Ma almeno, a quella data, se si ci dovesse rendere conto dell'impercorribilità dell'intero processo o di qualche sua pericolosa distorsione, si sarà ancora in tempo per introdurre correttivi e modificazioni all'impianto. Questo non toglie che l'assordante silenzio del Ministero dell'economia e delle sue tecnostrutture sia allo stato clamoroso e, se posso dire, Non c'entra il fatto che oggi - com'è stato detto - il ministro Tremonti sia a Bruxelles. Sono tre mesi che lo sollecitiamo, ed abbiamo potuto ascoltare in quest'Aula solo una discutibile disquisizione storico-filosofica sull'andamento delle politiche finanziarie e fiscali di questo Paese. Possibile, mi chiedo, che non si potessero simulare gli effetti per macroaggregati di spesa e di gettito tributario? Almeno come proiezioni di sfondo a cui parametrare le ipotesi delineate nel testo della legge delega, quale, proprio in carenza di quei riferimenti, ha dovuto mantenere un carattere di massima varietà di combinazioni ed opzioni aperte. Emerge qui, a mio parere, la contraddizione che si è cercato di mascherare, perché per promettere, come si è fatto, di tutto e di più a tutti è naturale che non si dovessero mettere in chiaro i numeri. Da questi, infatti, si sarebbe visto che il nuovo sistema, che è certamente più equo e rigoroso nella gestione delle risorse, anziché garantire rendite e premialità a gogò, richiede a tutti un *plus* di responsabilità e che si operi con determinazione ad ogni livello e latitudine per conseguire maggiore efficienza ed efficacia. maggioranza ad una maggiore prudenza perché risorse facili non ce ne saranno per nessuno. Piuttosto, ci saranno risorse appropriate per prestazioni e servizi di qualità in un sistema di regole che mette in mora incapacità e sprechi. Il che, almeno per noi, sarebbe già un gran bel risultato nell'interesse del Paese e dei conti pubblici. Per questo ci sarebbe piaciuto sentire parole chiare dal titolare del Dicastero dell'economia, a dissipare i timori di un appesantimento dei costi della pressione fiscale a regime (in merito ci sono nostri importanti emendamenti), sia anche perché temiamo che il suo riserbo nasconda una visione da *welfare* minimo e che sottintenda l'intenzione di proseguire nello scaricare il peso della quadratura dei conti su Regioni e Comuni, come si è fatto con l'ICI e il Patto di stabilità in questo avvio di legislatura, mettendo in grande difficoltà gli enti e le comunità territoriali che rispettano gli impegni, salvo poi derogare con compiacenza - nei casi di Catania e Roma che qui sono stati già ricordati - con buona pace di ogni criterio di uniformità e di equità di trattamento. dando atto delle cose positive che sono state introdotte nel lavoro di Commissione, mi soffermo su alcune sottolineature che vogliono essere critiche, problematiche e propositive. La prima, sotto il profilo fiscale. Continua a non convincerci, Ministro, il modello delle aliquote riservate sull'IRPEF per le Regioni e, soprattutto, la facoltà che viene data loro di intervenire con modifiche sulla base imponibile attraverso deduzioni, detrazioni e agevolazioni. È un problema molto delicato e complesso. Non so se ci si rende conto delle difficoltà che incontreranno, ad esempio, le imprese ad orientarsi in un ginepraio di questa natura quando ci saranno lavoratori che risiedono in vari Comuni, territori e, magari, in diverse Regioni. È così che si pensa di poter semplificare il fisco? Credo proprio di no. Capisco poi che si vogliano realizzare politiche di sostegno, per esempio, alle famiglie ed alle persone, ma si può agire con azioni positive senza ricorrere alla leva fiscale in questo caso, perché l'IRPEF è un tributo che ha una sua natura complessiva unitaria, progressiva. Disarticolarlo è un modo per snaturarlo con effetti regressivi e di probabile iniquità; e se anche oggi ci sono alcuni segni di queste distorsioni, vanno corretti visto che possiamo farlo. La seconda questione affronta un tema di ambiguità non risolta nella definizione compiuta dai LEP (livelli essenziali delle prestazioni) con riferimento all'assistenza. È un tema delicato anche questo. Non è chiaro come si intenda e soprattutto se si intende costruire gli standard di costi e fabbisogni e come si proceda a ripartire la copertura della spesa fra le Regioni e le funzioni riconosciute e finanziate ai Comuni. Da un lato, si dovrebbe pensare ad un sistema costruito in armonia con i LEA della sanità, ma poi la forfettizzazione della garanzia delle coperture finanziarie ai Comuni, parametrate sul meccanismo dell'80-20 (tra funzioni fondamentali coperte e quelle non fondamentali) sembrerebbe andare in direzione di soluzioni più semplificate e onnicomprensive. Ne discende il pericolo di una grande incertezza, soprattutto se consideriamo settori a grande rilevanza e intensità di prestazioni richieste, come asili nido o la non autosufficienza degli anziani o l'*handicap*; particolarmente, se si assume il tema di come costruire i meccanismi più appropriati per consolidare le realtà più avanzate e sostenere le situazioni più arretrate e conseguire per tappe intermedie il traguardo degli obiettivi di servizio considerati ottimali. Qui il testo della legge delega non ha previsto i meccanismi di traduzione operativa del processo di evoluzione dinamico e per questo noi riproporremo una serie di emendamenti che cercano di colmare questa lacuna. Da ultimo - signora Presidente, chiedo un minuto, se possibile, per completare un ragionamento - la questione delle funzioni dei Comuni. Qui torna il tema della disarticolazione rispetto al percorso della Carta delle autonomie. Questo delle funzioni dei Comuni era il punto più fragile della proposta originaria del Governo proprio perché troppo indeterminata. Nel lavoro di Commissione sono stati introdotti miglioramenti importanti: la garanzia della copertura del finanziamento per le funzioni trasferite, in modo da garantirne il normale funzionamento; una più precisa individuazione dei cespiti in grado di sostanziare l'autonomia finanziaria; la previsione di un meccanismo di garanzia nell'assegnazione delle risorse per la fase transitoria che si riassume nella formula 80-20. Ma è proprio qui che c'è un aspetto problematico, poco esplorato e per niente tranquillizzante. Per macro aggregati il sistema di finanziamento forfettario individuato può costituire una rassicurazione, e capisco che l'ANCI vi si sia riconosciuta, ma poi, come si incrocerà quello stesso criterio nel rapporto con il finanziamento che dovrà strutturarsi per costi standard e fabbisogni, stante l'enorme differenza di livelli, tipologie di servizi e prestazioni tra enti e geografie territoriali, in ragione di parametri

anche con successivi emendamenti. E allora, e concludo davvero, Presidente, più che agitare delle belle bandiere - come penso che forse qualche esponente della Lega si preparerà a fare - se si vuole costruire un impianto utile all'esigenza dei cittadini e dei territori, bisogna ripartire da questo testo così migliorato ed approfittare della discussione in quest'Aula, e del passaggio ulteriore che ci sarà alla Camera, per approfondire, simulare e specificare i contenuti di una delega che allo stato, seppur arricchita, resta ancora troppo ampia, discrezionale e farraginosa, con il pericolo di non conseguire gli obiettivi

penso che oggi sia un grande giorno, non solo per la Lega, ma per tutti i nostri militanti e per quegli uomini che sentono di avere un animo federalista.

con se stessi e nei confronti della società, e che vogliono operare nel mondo della politica per realizzare questi grandi cambiamenti, di cui ritengo la nostra società adesso abbia davvero tanto bisogno.

federalista: se, però, i tempi sono questi, sicuramente la carta di identità non me lo permetterà! Invece io mi auguro proprio di poter far parte, nel partito che rappresento e che mi onoro di rappresentare, del Senato di una Repubblica federale.

Grazie anch'io devo ringraziare il ministro Calderoli per il clima costruttivo che si è creato sia nelle Commissioni che in quest'Aula.

una riforma storica; credo che, dopo la Costituzione, sia quella più importante. Da parte nostra, sottolineo al Governo che, al di là del nostro posizionamento all'opposizione, non vi è alcun atteggiamento ipocrita e furbo. Abbiamo voluto collaborare e con la massima sincerità intendiamo contribuire fino alla fine dell'approvazione del

Il federalismo dei compromessi non serve, signor Ministro; noi dobbiamo portare avanti un federalismo convinto che possa giovare al bene del Paese.

in cui i livelli istituzionali - comunale, regionale e statale - sono l'uno contro l'altro armati. Il federalismo che noi sogniamo, lo Stato che noi sogniamo, è quello in cui c'è collaborazione tra i livelli di potere. Non è possibile

se il federalismo ha tardato è perché qualcuno voleva imporre determinati vantaggi per alcune parti del territorio. Il federalismo deve essere sì l'esaltazione delle diversità, signor Ministro, ma deve essere anche l'esaltazione della solidarietà massima

Bisogna orchestrare lo Stato in maniera diversa: le Regioni fondate nel 1970 sono state, sotto certi aspetti (e chi vi parla è stato per 11 anni un amministratore regionale), anche un fallimento nei riguardi delle autonomie locali, soffocando quella che è la Repubblica italiana nata sulle autonomie e sui municipi. Le Regioni oggi hanno usurpato tutto il settore dell'amministrazione attiva che deve competere ai Comuni. Ecco perché nella Carta delle autonomie - in cui dobbiamo fissarne i compiti - occorre

disegno dello Stato dei nostri Padri costituenti, in modo particolare della cultura cattolico-popolare, la celebriamo oggi proprio con questo tipo di federalismo che vogliamo portare avanti.

se non erro - 600 euro di trasferimento pro-abitante e a Padova 122. Certamente non li vogliamo togliere domani mattina, ma *in progress* dobbiamo far sì che ci sia

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, è stato detto da molti che la legge delega era partita in un modo e sembra arrivare in un altro. Francamente non sono sicuro che questa lettura sia del tutto corretta; penso che alcune delle differenze tra il testo uscito dalla Commissione e la proposta iniziale siano il frutto di una forse più attenta valutazione del Governo e della sua maggioranza, anche in seguito ad un'attenzione che noi abbiamo richiamato con le nostre proposte emendative svolgendo una funzione che è propria dell'opposizione soprattutto quando si determina un corretto rapporto nella dialettica parlamentare. Penso che quando il testo della legge é stato partorito dal Governo nelle sue fasi preliminari eravamo ancora sulla scia delle semplificazioni della campagna elettorale e dei messaggi semplici che dovevano far colpo,

Il primo cambiamento che vorrei sottolineare riguarda il contesto nel quale stiamo svolgendo questa nostra discussione, che è profondamente diverso da quelli che abbiamo conosciuto in altre occasioni quando abbiamo affrontato temi simili a questo. Penso alla *devolution* della stagione 2001-2006, alla riforma costituzionale di quella stessa stagione e poi, in conclusione, alla famosa riforma della legge elettorale chiamata in vario modo negativo, anch'essa frutto di quella stagione. Mi pare che ci sia una differenza nella discussione che noi stiamo sviluppando; questo sarà forse dovuto ad una sensibilità maggiore dei Ministri proponenti, che hanno registrato il totale fallimento della stagione 2001-2006 con la conseguente pesante

è una portata rilevante di carattere politico; stiamo tentando di rompere un tabù (non so se ci riusciremo) che finora ci ha impedito di realizzare importanti cambiamenti nel sistema di governo del Paese, di fare quelle riforme capaci di durare più di una legislatura, cioè più della legislatura che le vedeva approvate: ci lasciamo alle spalle questa tradizione tradizione non molto felice. È una sfida per la politica; penso che sia un modo attraverso il quale si possa riguadagnare quella fiducia perduta da parte dei cittadini nei confronti della politica. Il nostro punto di riferimento, nel merito della discussione, come è stato abbondantemente ricordato, è la riforma costituzionale del 2001, in particolare l'articolo 119. Come tutti hanno rammentato, siamo in grandissimo ritardo. Siamo appena all'inizio del 2009 e stiamo discutendo di una delega al Governo per l'attuazione di un precetto costituzionale che abbiamo introdotto già otto anni fa. anni fa. Inoltre, le tappe che caratterizzeranno la sua concreta attuazione richiederanno un arco temporale che consumerà quasi totalmente questa legislatura, arrivando fino al 2013. Dal 2001 al 2013 ci sono 12 anni; bisogna riflettere sul nostro modo di saper essere al passo con ciò che la società ci chiede. abbiamo letto e sentito tesi e discorsi che hanno richiamato noi legislatori ad una riflessione su come si sia esaurita la spinta che originò la riforma del Titolo V e sul fatto che forse siamo in presenza di un ripensamento centralista nella funzione di governo dello Stato. Personalmente considero sbagliate questi tesi e credo che sarebbe un danno per il Paese e per la stessa democrazia immaginare un salto all'indietro. Il giudizio che dobbiamo dare complessivamente sull'esercizio del governo esercitato da Regioni, Comuni e Province è nell'insieme positivo, sia per gli effetti che ha prodotto, sia per il sistema di democrazia che cresce. Non credo che possiamo tornare indietro: l'autogoverno e il federalismo ad esso collegato è modernità; il centralismo è passato e sarebbe un salto indietro grave se dovessimo compierlo. Si discute ancora se questa è una riforma principalmente incentrata sulle risorse. Abbiamo parlato molto, nella fase preparatoria della discussione in Commissione, su chi ci guadagnerà e chi ci rimetterà, ovviamente rispetto alla situazione storicamente consolidatasi. Attualmente - per citare alcuni dati di riferimento - il 18 per cento dei pagamenti del bilancio dello Stato sono trasferimenti al sistema locale per cento della spesa centrale ha un impatto regionale. Questo, qualche tempo fa, portava qualche illustre costituzionalista, ma più economista, a dire che di fatto il federalismo in Italia è già in atto. non sono d'accordo, perché se il 78 per cento della spesa del bilancio dello Stato ha un impatto regionale, tutto viene deciso al centro e ciò che conta è il luogo nel quale vengono prese le decisioni che determinano la cosiddetta spesa.

quasi completamente abbandonate nel testo. Non credo però siano state abbandonate nelle intenzioni, e questa è la ragione per la quale abbiamo un giudizio sospeso fino alla fine.

livello di sviluppo tra le diverse aree del Paese davvero profondo. La Costituzione ha giustamente previsto all'articolo 119 come si deve tener conto di queste differenze e infatti i principi della delega di cui discutiamo si articolano con l'obiettivo di realizzare un federalismo che abbiamo definito contemporaneamente solidale e responsabile. Come è evidente, la solidarietà è un principio fondamentale di coesione di una comunità nazionale, ma è tanto più sentita quanto più esiste il bisogno. la solidarietà viene richiamata perché questo è un Paese che ha ancora troppe differenze. Sappiamo che l'Italia del 2009 per essere coesa ha l'obiettivo di ridurre le differenze di sviluppo che ha registrato finora. questo dato strutturale tuttavia non può essere invocato, come è stato fatto finora per troppo tempo, per contrastare un'idea di federalismo e quindi di autogoverno.

della perequazione verticale. Lo Stato, e solo lo Stato centrale, deve esercitare questo ruolo perequativo. In conclusione, penso che il Governo e la maggioranza hanno una responsabilità importante, politica e di merito. Se questo atteggiamento prosegue, mantenendo il clima di attenzione e confronto positivo fra maggioranza e opposizione registrato in Commissione, sarà un bene per questo provvedimento ma anche per gli altri importanti provvedimenti di riforma che ci attendono in questa legislatura. Per questa ragione rivolgo un invito a valutare con apertura le nostre ulteriori proposte emendative, come ha sottolineato efficacemente il nostro relatore di minoranza.

Grazie e riguardano innanzi tutto il tema del rapporto fra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale, che non è una questione accademica né teorica. L'unico esempio vivente di federalismo istituzionale e fiscale esistente nel nostro Paese è quello disegnato dal sistema delle specialità, dagli Statuti speciali che, come noto, sono norme costituzionali. Possono piacere, possono non piacere, possono essere considerati dei privilegi e possono non esserlo considerati. Vi è forse anche l'esigenza del superamento degli Statuti speciali. Tutte argomentazioni nobili, queste, ma c'è un piccolo, trascurabile dettaglio dal quale non si può prescindere: sono norme costituzionali che non possono essere modificate unilateralmente dallo Stato con legge ordinaria. é - e così è - la prima questione che poniamo è che vi sono almeno tre disposizioni della delega, così come modificate in Commissione, che sono in aperto contrasto con gli Statuti speciali, in modo particolare con quello della Regione siciliana. La prima disposizione è l'articolo 14 che riguarda la disciplina, la istituzione ed il funzionamento delle Città metropolitane. Questa è una materia riservata dall'articolo 14, comma 1, lettera *o)* dello Statuto siciliano alla competenza esclusiva della Regione. Non può intervenire lo Stato su questa materia. Ripeto, piaccia o non piaccia, io non sto ad esprimere qui una valutazione di merito. quella che in maniera molto originale avete definito la perequazione infrastrutturale, disciplinata dall'articolo 21 della delega, in cui voi dite due cose: la prima è che nella fase di prima applicazione del federalismo fiscale si istituisce una cabina di regia, composta da quattro Ministri, i quali devono fare una ricognizione del fabbisogno infrastrutturale

prevede per lo sviluppo economico, la coesione sociale e la eliminazione delle differenze territoriali, soprattutto con riferimento

in deroga ritengo a tutte le disposizioni riguardanti la programmazione delle opere pubbliche (quindi il CIPE e tutti gli altri organi di programmazione statale e regionale) sia uniformata al criterio della premialità rispetto a chi, in tempi più rapidi, riesce ad allinearsi al criterio del costo standard e quindi a criteri di efficienza. Se così

al comma 1 dispone: «Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici» «Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale». non è complementare o aggiuntiva rispetto alla norma costituzionale contenuta nello Statuto, che disciplina le modalità attraverso le quali lo Stato interviene con il contributo di solidarietà nazionale nella Regione siciliana per la realizzazione di opere a compensazione del minor reddito da lavoro, quindi non c'entra neanche la capacità fiscale per abitante, è evidente che questa disposizione cozza, in maniera chiara, con con i principi che regolano le autonomie speciali e nel caso di specie quello della Regione siciliana. La terza disposizione, signor Ministro, è quella che riguarda l'articolo 25 del testo della delega che reca disposizioni, in forza delle quali bisogna coordinare la finanza dello Stato, e segnatamente quella introdotta nella delega fiscale, con la finanza delle Regioni a Statuto speciale. Al di là della enunciazione di una serie di principi che fanno riferimento alle norme statutarie, alle Commissioni paritetiche e quant'altro ed alle norme di attuazione, voi dite sgrezzato da principi aulici e condivisibili quali quelli contenuti negli Statuti ed anche in quello della Regione siciliana - che ciò che si applica, comunque, nella definizione del rapporto finanziario tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale, quindi tra lo Stato e la Regione siciliana, è il principio del costo standard e del superamento del principio della spesa storica. Condivido, in linea generale, l'applicazione del principio del superamento della spesa storica, ma certamente questo non sfugge alla regola costituzionale, sancita

È quella la sede in cui voi avete il diritto-dovere di intervenire per cambiare il meccanismo di finanziamento.

anche dal vostro punto di vista e dalla vostra prospettiva federalista uno dei cardini e cioè la circostanza che tutta la materia, così come disciplinata anche per le Regioni a Statuto ordinario dalla nuova formulazione dell'articolo 114, è oggetto di negoziazione, tant'è vero che voi la prevedete, secondo me illegittimamente, nella Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si sostituisce al Parlamento nella definizione dei criteri in ordine alla perequazione, per stabilire l'entità delle risorse e per controllare che queste vengano effettivamente gestite al meglio. Quindi, questa è la prima questione che ci permettiamo di sottoporvi, anche perché

che per queste ultime la materia dell'armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica, essendo oggetto di legislazione concorrente, ha bisogno di princìpi fondamentali (che in questa sede noi dovremmo fissare, e che abbiamo fissato in maniera generica), mentre per le Regioni a Statuto speciale non vi è bisogno che lo Stato intervenga fissando i princìpi fondamentali perché questi le Regioni possono ricavarli dai princìpi fondamentali di riforma economica e sociale che riguardano il nostro Paese, e lo fanno autonomamente nel momento in cui legiferano in materia tributaria e fiscale. Si tratta di una questione centrale dal nostro punto di vista, su cui si misura, per quello che a voi può interessare, la nostra posizione in merito al voto finale su questo provvedimento. La seconda questione, signor Ministro, riguarda la vicenda delle funzioni. È noto che il testo sul federalismo fiscale sconta il limite genetico della confusione relativa al riparto di competenze tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie, così come introdotto dall'articolo 117 della Costituzione, a seguito della riforma entrata in vigore nel 2001, votata, lo ricordo, a maggioranza dall'allora Governo di centrosinistra.

le opere infrastrutturali, che sono anch'esse oggetto di legislazione concorrente e che hanno scontato il limite di sentenze della Corte costituzionale, ad esempio su una legge importante e strategica per il nostro Paese quale è stata la legge obiettivo, approvata nella legislatura 2001-2006.

dal quarto comma, ma anche per quanto riguarda le materie concorrenti; quindi, per tutte le materie indicate al terzo comma dell'articolo 117, le Regioni hanno una potestà regolamentare esclusiva.

alla Corte costituzionale il compito di dare un'interpretazione del nuovo assetto dei poteri che fosse coerente con le esigenze di sviluppo di un Paese civile. Oggi, quindi, ci troviamo con questo limite che comporta che, dal nostro punto di vista, è difficile (ed è un tema che va chiarito) poter procedere al riparto delle risorse, e quindi dell'autonomia impositiva correlata, se non si identificano con chiarezza i livelli essenziali delle prestazioni (ad esempio (ad esempio di quelle indicate alla lettera *m)* dell'articolo 117). Sono livelli che dalla nostra prospettiva noi riteniamo siano ancora essenziali, ancorché voi abbiate scelto un'altra strada, e che dovrebbero essere completamente finanziati dallo Stato.

non è chiarita (o sembra essere chiarita e abbandonata) la scelta, che ci appariva più logica, della soppressione delle Province. Invece oggi si attribuiscono alle Province una serie di si conferma pertanto la loro utilità: ne prendiamo atto, ma che nessuno venga poi a dire che su questo punto vi è un'altra posizione. Contemporaneamente, si sovrappongono alle Province le aree metropolitane senza definirne contenuti e funzioni.

ma è giusto che nella definizione del concetto di costo standard non entri il costo della inefficienza delle pubbliche amministrazioni, così come non è giusto che non vi entri la determinazione delle diseguaglianze territoriali che determinano aree di mercato diverse e costi diversi delle prestazioni. In caso contrario, questo differenziale viene caricato sulla fiscalità generale, in particolar modo sulla fiscalità del Mezzogiorno d'Italia e in particolar modo sulle addizionali IRPEF necessarie a coprire questo tipo di risorse.

Non c'è traccia, nel provvedimento, di chi e di come si faccia carico del debito pubblico. Noi riteniamo che questo compito sia in capo allo Stato e, se così è, il livello dell'imposizione fiscale statale chiaramente non può scendere e non vi è certezza sui conti e sulla sostenibilità economica del provvedimento che stiamo esaminando, salvo il fatto che non accettiamo accettiamo e non dobbiamo accettare e dare per scontato che vi sarà un aumento dell'imposizione fiscale locale vista l'ampia autonomia...

stesso modo, non si può sottrarre al Parlamento il compito di legiferare e di controllare il fondo perequativo previsto dall'articolo 119 della Costituzione. In questo modo, si sposta l'asse della democrazia in un'altra direzione. Su tali questioni siamo pronti al confronto, e se ci sarà disponibilità, non abbiamo difficoltà a confermare o a cambiare opinione rispetto a quella tenuta in Commissione. Altrimenti, voteremo contro

Ho fatto questo riferimento per inserire una valutazione che altri colleghi in Aula hanno ripreso - in particolare il senatore Morando - a proposito del Titolo

Grazie

spingere il piede sull'acceleratore ed impostare nuovamente una riforma globale costituzionale decidendo piuttosto di intraprendere in senso pragmatico - un merito che va riconosciuto indubbiamente al ministro Calderoli - un percorsodi riforma che potesse trovare una convergenza

virtuoso, di crescere in senso organico e di avvicinarsi. Credo che l'aspetto dei costi standard, che prevede però l'assoluta certezza di garantire il livello dei servizi a tutti i cittadini italiani, ma al tempo stesso di creare quell'elemento

l'ultimo elemento, che può cogliere il nostro Paese per crescere insieme e per far sì che le zone meno che le zone meno efficienti del nostro Paese possano diventarlo emulando quelle che lo sono maggiormente. Naturalmente la mia non è una visione utopistica; è una convinzione concreta, che nasce anche dall'esperienza di amministratore che ho potuto maturare in questi anni.

(se nei confronti della Corte costituzionale si può avanzare qualche critica) nel contrastare l'attuazione della legge obiettivo, che, proprio in un periodo di recessione come questo, in cui c'è l'assoluta necessità di riprendere gli investimenti nelle opere pubbliche, avrebbe potuto essere uno strumento estremamente utile per agevolare e per promuovere gli investimenti infrastrutturali.

un aspetto che non ci possiamo più permettere; è un costo dell'inefficienza della macchina pubblica che non possiamo più sopportare. C'è pertanto l'assoluta necessità di rivedere Concordo con il collega D'Alia: le materie sono quelle del turismo e delle infrastrutture. Si prenda un tema come quello dell'energia, che è oggi una materia concorrente tra lo Stato e le Regioni; onestamente, credo che questo non sia più possibile. Le Regioni sono d'accordo a rivedere l'attribuzione di queste materie. Il progetto di riforma costituzionale della devoluzione aveva al suo interno questi elementi e queste definizioni.

l'importante e sempre puntuale presenza ai lavori in Commissione, per la disponibilità ad un confronto costruttivo tra maggioranza e minoranza e per la disponibilità nei confronti degli alti livelli istituzionali auditi, come anche nei confronti delle varie rappresentanze del mondo economico. Complimenti, quindi, ministro Umberto Bossi, e complimenti, ministro Roberto Calderoli. Un notevole apprezzamento va poi al lavoro sempre preciso e chiaro del relatore, il senatore Azzollini, e dei Presidenti delle Commissioni come anche al contributo positivo contenuto nell'intervento di questa mattina del relatore di minoranza, senatore Walter Vitali. Di grande rilievo ritengo siano, inoltre, da considerarsi i molti interventi parlamentari svolti in Commissione, sia di maggioranza che di minoranza, dai quali trasparivano per lo più aspetti propositivi e lodevole capacità di uscire dai rispettivi schieramenti e di evidenziare quanto di buono è contenuto nel provvedimento in oggetto. Ma sorprende e dispiace, lo dico senza alcuna nota polemica, dover rilevare come le tante positività espresse nella riservata Aula delle Commissioni quasi svaniscano in alcuni interventi ascoltati oggi nella più pubblica Aula del Senato. Di grande importanza inoltre sono state le molteplici audizioni che in Senato, nelle Commissioni 1a, 5a e 6a riunite si sono succedute, oltre a quelle svolte nella Commissione parlamentare per le questioni regionali. Lo stesso Governo in più occasioni ne ha sottolineato, del resto, l'utilità e il positivo contributo. Infine, non può essere dimenticato l'intervento del Presidente della Repubblica che sentenzia come l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ovvero del federalismo fiscale, sia una necessità. Colleghi, spesso ci ritroviamo in quest'Aula ad esaminare provvedimenti che sono buoni, altre volte ci troviamo ad esaminare provvedimenti che sono opportuni ed altre ancora provvedimenti invece urgenti e necessari. Questo provvedimento, non perché lo diciamo noi,

Risulta quindi essere buono, opportuno, necessario ed urgente. Il Paese sta per essere messo, quindi, nei binari giusti. Purtroppo, però, lo si sta facendo in zona Cesarini, incalzati da esigenze di bilancio per le famiglie, le aziende, le istituzioni. Guai quindi a non procedere, a perdere altro tempo, che ormai non c'è più. Non a caso, infatti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime un parere positivo sui principi contenuti nel provvedimento in esame. In effetti, sono proprio i valori contenuti nel testo legislativo in esame a fare da cordone ombelicale tra il Paese e le istituzioni. Sono i valori a legare le varie Nazioni, i popoli, i cittadini contribuenti ai loro rappresentanti, oggi sempre troppo distanti dal territorio. Valori e principi quali l'autonomia e la responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo; quali il principio di territorialità dell'imposta (quindi, avremo la possibilità di reperire i fondi per finanziare le competenze in modo autonomo da parte delle Regioni e degli altri enti locali); quali il principio innovativo che prevede il superamento del criteri della spesa storica a favore della spesa standard. l'esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto (quindi, no alle doppie tasse, nel pieno rispetto dei valori contenuti nel famoso Statuto del contribuente). Principi e valori quali la correlazione tra prelievo fiscale e benefici che favorirà un miglioramento della responsabilità amministrativa. Valori e principi quali quello per cui si premieranno i comportamenti virtuosi ed efficienti e si puniranno le incapacità, nel pieno rispetto dei criteri di meritocrazia e di buonsenso. Valori e principi quali la semplificazione del sistema tributario, con la riduzione degli adempimenti a carico del contribuente: basta quindi pagare per pagare poi le tasse; stop alla burocrazia, divenuta una tassa sulle tasse, che poi si devono andare a pagare. Principi e valori quali la razionalità e la coerenza dei tributi o quali la riduzione dell'imposizione fiscale statale la riduzione dell'imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed altri enti locali, perché, come evidenziato nel provvedimento, il saldo in positivo, ai vari livelli di governo, deve determinare una riduzione complessiva della pressione

attraverso un emendamento, poi recepito direttamente nel testo, all'articolo 15: più precisamente si prevede il totale fallimento politico di un amministratore incapace che manda in dissesto l'istituzione da lui rappresentata. In altre parole,

Sono quindi questi i valori e i criteri di buonsenso, già condivisi tra l'altro nella Carta costituzionale, ma oggi metabolizzati nel DNA delle più importanti e meritevoli culture del nostro Paese. sono questi i valori che consentiranno l'andare "a dama" del federalismo fiscale, in considerazione del fatto che ne rappresentano l'essenza; e tanto più urgente è questo risultato, quanto più è vero che stiamo subendo una crisi di vaste dimensioni. La crisi attuale, infatti, unita all'imponente debito pubblico e ai sovradimensionati costi dello Stato, non deve mettere paura nell'imboccare la via del cambiamento, anzi, anzi, deve essere un acceleratore, un motivo in più per fare in fretta, per non rimandare o sprecare tempo ulteriore. E allora, avanti tutta e, direi, avanti tutta e tutti insieme, maggioranza e minoranza, anche perché finora si è speso tanto e male, mentre diventa obbligo imperativo diminuire la spesa e soprattutto migliorarla, in modo da consentire la riduzione, in un futuro quanto più prossimo, della pressione fiscale, avendo garantito tra l'altro che si eviti ogni duplicazione di funzioni. Colleghi, provengo dal mondo dell'impresa, ma quando la mia o le altre realtà economiche sono in difficoltà, non ricercano qualche contributo che che arrivi come la manna dall'alto, qualche sussidio risolutore, ma si sforzano semplicemente di diventare più competitive sul mercato. Lo stesso deve valere per l'"azienda Paese" che non può pensare di andare avanti cercando di inventare ogni volta qualche trucco, dovendo invece semplicemente diventare più competitiva: tanto più c'è competizione tra Regioni quanto più la gara virtuosa a chi è migliore porterà al miglioramento dell'"azienda Paese" e alla vittoria del modello federale. Il federalismo fiscale costituisce, quindi, uno strumento di politica economica capace di rendere più efficienti, trasparenti e competitive le pubbliche amministrazioni, garantendo così maggiore qualità di servizi, con costi evidentemente minori. Non solo: il federalismo fiscale consentirà di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di servizi. Oggi, al contrario, si sono impiegate quantità incredibili di denaro, con il risultato altrettanto incredibile di non avere risultati omogenei di servizi nel territorio. Quindi, l'obiettivo sarà quello di abbassare la spesa corrente, qualificando la spesa stessa e razionalizzandola, responsabilizzando l'operato degli amministratori pubblici consentendo così un rientro nei costi dello Stato e la possibilità di incrementare la spesa per investimenti in conto capitale, capaci - questi solo - di creare vero Tale strada, del resto, è stata imboccata nelle politiche macroeconomiche scelte dal Governo attuale, ma alle politiche fiscali e macroeconomiche occorre affiancare - appunto - questo federalismo fiscale, altrimenti il *cocktail* medicamentoso certamente non riuscirà a guarire il nostro Paese. Si tratta di un *cocktail* che per il Sud dovrà passare anche attraverso un'azione di bonifica da mafie e malavita;

Tutto ciò sarà possibile solo - ripeto - se diverrà realtà questo federalismo fiscale. Con evidente entusiasmo, quindi, invito il Governo a proseguire perché questa è la strada giusta, quella che vuole percorrere la stragrande maggioranza del Paese. Dunque, avanti tutta e tutti insieme, signori Ministri. Buon lavoro e diamo il benvenuto al federalismo fiscale!

Il radicamento nel territorio delle politiche per le persone, per le famiglie e per le imprese, la valorizzazione delle specificità, delle diversità e delle energie locali, la valorizzazione delle autonomie locali nel quadro dell'unitarietà dello Stato sono assi culturali di riferimento delle nostre politiche. Non a caso la riforma del Titolo V della Costituzione è stata voluta ed approvata dal centrosinistra. conveniamo sull'opportunità di fare delle modifiche, ma è indubbio che sia stata una scelta fortemente autonomista e - ricordiamo - convalidata da un *referendum* confermativo. Io ho maturato la mia esperienza politica prevalentemente in Comune e nella Regione Emilia Romagna, la quale storicamente ha puntato ad una forte valorizzazione delle autonomie locali come perno dello sviluppo economico e della qualità sociale.

investimenti sulla formazione e sull'istruzione, sviluppo economico e quindi collegamento e sostegno ai suoi attori (imprese ed altro), occupazione (anche femminile),

Da queste considerazioni e nel doveroso rispetto del complesso del testo costituzionale, sia nei princìpi fondamentali sia nei suoi articoli 114, 117, 118 e 119, e 119, che non configura un regionalismo, cioè uno Stato federale basato sulle Regioni, ma una vera valorizzazione delle autonomie locali,

federalismo è entrato nel linguaggio politico e nel linguaggio corrente per volontà e per capacità della Lega. Ora si tratta, a mio avviso, di un uso improprio, a fronte di un testo di legge che si è fortemente allontanato dal provvedimento della Lombardia che configurava un regionalismo spinto, egoistico e con la perequazione orizzontale. Oggi questo testo, che era stato assunto dal Popolo della Libertà nel proprio programma elettorale, è stato superato già dal testo del Governo che

una competizione selvaggia e una sorta di autarchia (tutti elementi di cui questo Paese non ha assolutamente bisogno), occorre individuare un forte ed innovato ruolo dello Stato. Occorrono norme generali, chiare e senza sovrapposizioni e princìpi fondamentali. Infatti, norme generali e princìpi fondamentali sono i binari necessari per la legislazione regionale nelle materie concorrenti e per le funzioni amministrative di tutti i soggetti locali. poi definire le funzioni fondamentali di Comuni e Province, i livelli essenziali delle prestazioni, la definizione dei costi standard, i fabbisogni ottimali e l'avvicinamento progressivo a quei fabbisogni ottimali, al fine di garantire i diritti fondamentali dei cittadini. Sono tutti questi elementi caratterizzanti dell'identità dello Stato unitario e del sistema delle autonomie locali. locali. È un impianto complesso e difficile, ma d'altra parte - lo sanno benissimo i rappresentanti del Governo e noi del Partito Democratico - per fare delle riforme occorre uno sguardo lungo e obiettivi alti. Il disegno di legge che discutiamo contiene dei miglioramenti significativi che sono derivati da un lavoro lungo ed impegnativo in Commissione e nel Comitato ristretto. Sottolineo la doverosa attenzione e le aperture proposte dai rappresentanti del Governo e della maggioranza. Si è costituito un dialogo vero doverosamente collocato nelle sedi istituzionali - e importante per le riforme, anche se durante questo dialogo, purtroppo più volte ci sono stati interventi del Presidente del Consiglio che miravano a negare e a ostacolare questa possibilità. Sono migliorate parti significative del testo. Ne cito una per tutte: il principio della territorialità che è stato ben definito. Vi sono però ancora contraddizioni e parti fortemente carenti: il senatore Vitali è stato molto preciso nell'elencarle.

dove tutti conveniamo che ci sono sovrapposizioni, duplicazioni di competenze e frammentazioni. È un'incongruenza gravissima del disegno di legge, che ne mina alle fondamenta la capacità di innovazione e di riforma, risultando fortemente conservativo rispetto alla situazione esistente. D'altra parte, è abbastanza incongruente che siano definite prima le risorse che le funzioni. Secondo punto: manca la riforma costituzionale con il superamento del bicameralismo perfetto e l'istituzione di una Camera delle Regioni e delle autonomie locali. Il fatto che nel testo sia molto spesso richiamata la necessità preventiva di un'intesa in Conferenza unificata segnala, da un lato, questa carenza della Camera delle Autonomie, e determina anche un forte svuotamento Terzo punto: la mancanza di dati e di proiezioni credibili su quello che si verrà a definire quando queste norme troveranno attuazione. L'ultimo punto del mio intervento riguarda la relazione tra il federalismo fiscale e la crisi economica. Siamo di fronte ad una crisi economica profonda e strutturale. I dati sul prodotto interno lordo e sui consumi e, conseguentemente, sul calo delle entrate e sull'esplosione del debito pubblico, sono davanti tutti noi. Noi vogliamo e possiamo uscire da questa crisi in avanti, così come ha autorevolmente proposto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con un Paese in cui ci siano più opportunità e più uguaglianze. Sono, quindi, necessarie per queste uscite in avanti delle innovazioni forti, delle scelte e delle priorità ben individuate, caratteri tutti che non vedo in questo disegno di legge delega che sembra dare tutto a tutti, in una logica più di rassicurazione che di scelte e di determinazione in avanti del futuro del Paese.

produrre sviluppo economico, coesione sociale e per dare più opportunità alle persone, alle imprese e al Paese tutto; se credono che ci sia un'opportunità di sostenere le azioni dello sviluppo locale nel contesto della globalizzazione, così come hanno fatto nel passato importanti Regioni, che sono una punta avanzata in tutto il sistema italiano e anche nel contesto europeo. Personalmente penso che questa sia una strada giusta. Sono convinta che due volani fondamentali per l'uscita dalla crisi siano, oltre al contesto internazionale, da un lato, un forte investimento nel nostro Paese sull'istruzione, sui saperi, sulla ricerca e sulle competenze delle persone e, dall'altro, sulla sulla valorizzazione dello sviluppo locale. Parlo di valorizzazione delle intelligenze dei giovani, delle donne, delle opportunità e delle straordinarie risorse che ci sono nei nostri territori e che nel nostro Paese non sono sufficientemente valorizzate. Dobbiamo considerare tutto ciò non come un ragionamento marginale, ma al contrario come la strategia fondamentale individuata dall'Unione europea. Credo, in sostanza, che il fatto che si evitino sprechi, il fatto che si evitino delle rivendicazioni di risorse continue e degli "scaricabarile" di responsabilità sia un'opportunità positiva e straordinaria nel nostro Paese. Concludo dicendo che chi, invece, non è convinto di ciò, chi pensa il contrario e cioè che ci siano dei rischi importanti per l'economia nell'aumentare le responsabilità delle autonomie locali nel prelievo e nella spesa, chi pensa, come si sta praticando oggi da parte di questo Governo,

Signora Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte al difficile compito di razionalizzare o, meglio, di modernizzare il sistema di redistribuzione delle risorse all'interno del nostro Paese. Il federalismo fiscale rappresenta una tappa fondamentale verso quella trasformazione così necessaria alla modifica dell'organizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato. Si parte da un dato certo ed incontrovertibile: così com'è attualmente dimensionata la macchina statale ha dimostrato di non poter funzionare, dando il fianco allo spreco di illimitate risorse economiche per interventi di sostegno, spesso *una* *tantum*, a porzioni di territorio che per nulla hanno usufruito di tali benefìci. I dati sulla ricchezza nazionale dimostrano ampiamente questa situazione. Dico, quindi, sì e al disegno di legge che porta il nome del collega Calderoli, che ha messo competenza e entusiasmo nel provvedimento che oggi discutiamo. Abbiamo dibattuto a lungo in questi anni di sussidiarietà, di valorizzazione delle autonomie locali, di responsabilizzazione dei vertici degli apparati periferici dello Stato e degli enti territoriali; è arrivato, dunque, il momento di dare corpo alle nostre idee e con convinzione, insieme ai colleghi del Gruppo PdL, aderisco a questo progetto. Pongo, però, alcune riflessioni su un tema a me caro quale quello del diritto alla salute del cittadino che trova già ampia tutela nell'attuale testo in esame, ma che i successivi adempimenti normativi (decreti legislativi) dovranno via via sempre più salvaguardare. Mi riferisco alla pari dignità nel diritto di tutti i cittadini di ricorrere alle prestazioni sanitarie. L'inopportuna riforma del Titolo V della Carta costituzionale dell'anno 2000, la cosiddetta riforma Bassanini, ha di fatto sancito la fine del modello socio-assistenziale che ha caratterizzato l'unitarietà dell'offerta sanitaria del nostro Paese, mediante il trasferimento di tutti i poteri alle Regioni e favorendo, nei fatti, la nascita di una somma di sistemi sanitari regionali con un alto grado di diseguaglianza. Il riordino della sanità non è fatto solo di tagli di posti letto e/o di prestazioni varie; anzi, spesso la riduzione di offerta comporta un aumento dei costi assistenziali. Le cronache a volte tragiche di questi ultimi anni e i risultati dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale del Senato, di cui mi onoro di aver fatto parte nella scorsa legislatura, hanno mostrato inequivocabilmente una Italia divisa in due, dove il Nord si caratterizza per un'offerta sanitaria di eccellenza e il Sud per un sistema sanitario di sicuro non riferito a certe alte professionalità che vi operano, la cui organizzazione e struttura di riferimento presenta lacune spesso incolmabili. Questo evidenzia che l'equazione risorse finanziarie uguale qualità delle prestazioni non è affatto dimostrata; anzi, l'attuale sistema di finanziamento della spesa sanitaria ha di fatto creato due sistemi distinti che marciano a velocità differenti. Non più costo storico - ed è giusto - ma standardizzazione dei costi; è questo il principio regolatore dei flussi finanziari a disposizione delle Regioni per far fronte alle spese della sanità nazionale. Non più fondi trasferiti ma risorse proprie, con le quali le Regioni più virtuose sapranno ancor più migliorare i loro standard socio-assistenziali, mentre le altre avranno il dovere di mettersi alla pari con le prime, ma senza terremoti. legge in esame prevede espressamente all'articolo 7 la presenza di un fondo perequativo che assicurerà alle Regioni, non in grado di prevedere adeguati fabbisogni finanziari sulla base della ricchezza per singolo cittadino, risorse aggiuntive tali «da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni». D'altro canto, in materia sanitaria, il processo di responsabilizzazione delle Regioni era già iniziato da tempo, con la netta distinzione tra fabbisogno e spesa storica. Vorrei ricordare che l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 già segnava il passaggio ad un sistema di finanziamento della spesa sanitaria non più agganciato alla spesa storica (in cui lo Stato è intervenuto ripianando la spesa a piè di lista), bensì ad un livello di fabbisogno valutato come rapporto ottimale rispetto al PIL. Ne consegue che, in campo sanitario, Governo e Regioni avevano già maturato la scelta di superare il concetto di spesa storica consolidatasi nelle singole realtà regionali e di individuare un livello di fabbisogno predefinito al cui finanziamento concorre lo Stato nel rispetto della piena erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Con l'accordo del 2001 viene inoltre sancito un ulteriore principio che nel tempo si è rivelato di assoluta efficacia, cioè il fatto che, nell'assegnazione annuale delle risorse alle singole Regioni, una quota di esse (inizialmente fissata al 4-5 per cento e poi viene considerata premiale e, quindi, effettivamente erogata solo a seguito di una verifica annuale che attiene sia al mantenimento dell'equilibrio di bilancio che all'erogazione effettiva dei livelli essenziali di assistenza. Da ultimo, anche il nuovo Patto sulla salute pone in risalto la volontà di dare certezza di risorse per il Servizio sanitario nazionale. La vigente legislazione, in tema di riparto delle perdite del Servizio sanitario nazionale, inserita nel più ampio contesto normativo del federalismo fiscale, prevede che a ciascun livello istituzionale venga attribuita la responsabilità di spesa derivante dalle rispettive potestà decisionali. Per quanto riguarda i provvedimenti normativi di ripiano dei disavanzi intervenuti nel corso degli ultimi anni (con riferimento alle leggi di ripiano per gli anni 2001-2005), si è progressivamente passati da una confermata tendenza a spalmare fra tutte le Regioni le risorse destinate al ripiano di disavanzi fino alla odierna impostazione, soprattutto a seguito del Patto per la salute 2006, che prevede di non riconoscere aprioristicamente risorse a piè di lista in favore di tutte le Regioni, ma di attribuire le stesse in funzione del concorso da parte delle Regioni nella formazione dei disavanzi. Per quanto concerne l'esigenza di prevenire il formarsi di nuovi disavanzi, a partire dal 2005 sono stati introdotti meccanismi di deterrenza, fondamentalmente costituiti dall'obbligo, in caso di disavanzo non autonomamente coperto dalla Regione, di incrementare automaticamente, nella Regione interessata, fino al livello massimo, le misure fiscali regionali di interesse sanitario (addizionale IRPEF e maggiorazione IRAP). I nuovi rapporti finanziari Stato-Regioni, all'interno dei quali risulta predominante la tematica del finanziamento della spesa sanitaria, saranno disciplinati dal provvedimento legislativo che sostituirà il decreto legislativo n. 56 del 2000. Ed è qui che richiamo l'attenzione dei colleghi e del Presidente. I principi assolutamente condivisibili dettati dall'attuale testo normativo dovranno trovare concreta attuazione nei successivi e specifici decreti legislativi, che dovranno tener conto inesorabilmente della pari dignità dei cittadini italiani grazie a tutto pur se legittimamente erogato, in termini di organizzazione, a livello regionale. Sarebbe, come oggi è, eticamente e politicamente scorretto che una persona possa ritenersi fortunata se nasce in una Regione, sfortunata se nasce in un'altra. Sarà anche specifico compito dei successivi decreti legislativi quello, tra gli altri, dell'istituzione del fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito IVA assegnata per le spese per i livelli essenziali delle prestazioni, nonché da una quota del gettito del tributo regionale. Secondo i dati forniti dal *Welfare*, la disciplina sul federalismo fiscale fisserà la definizione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale e dei singoli sistemi sanitari regionali ai costi standard. A tal proposito, lo stesso Ministero del *welfare* ha preparato una simulazione dalla quale si rileva che applicando a tutte le Regioni i costi registrati nelle due amministrazioni più efficienti, individuate nelle regioni Lombardia e Veneto (costi standard), si prospetterebbe un teorico risparmio di 4,5 miliardi di euro l'anno. Nel modello si introducono criteri di pesatura delle varie popolazioni regionali per fasce di età; tale dato si riduce in maniera più o meno rilevante a secondo dei criteri utilizzati. I finanziamenti che si renderebbero disponibili a seguito di tale risparmio potrebbero essere mantenuti nel settore sanitario, promuovendo politiche di razionalizzazione e qualificazione dei servizi, in modo da orientare il Servizio sanitario nazionale su obiettivi di efficienza, qualità e sostenibilità. Ciò appare compatibile con la prospettiva connessa all'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare quelle connesse alla informatizzazione, all'automazione e alla telemedicina: per cento della spesa sarà assorbita dai servizi sociosanitari e assistenziali di tipo territoriale, in grado di assicurare la «presa in carico» dei singoli e delle fasce di popolazione a rischio di cronicità. Il nuovo Patto sulla salute 2010-2012 tra Stato e Regioni, potrà garantire che nel finanziamento assicurato sia prevista una quota calcolata in base al numero degli abitanti di ciascuna Regione e al costo per abitante delle Regioni assunte come standard; e una quota aggiuntiva ma decrescente che per un certo periodo di tempo sostenga le Regioni nell'adeguamento dalla spesa storica al costo standard. Tutto questo per favorire e garantire un livello di un livello di eccellenza e di qualità a tutela del servizio dei cittadini e di uno Stato efficiente che faccia fino in fondo il proprio dovere nel rispetto dell'articolo 32 della nostra Carta costituzionale.

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Ministro, siamo giunti a questo appuntamento muovendoci lungo un percorso serio, rigoroso, non certo ostruzionistico da parte del nostro Gruppo; un percorso che ha visto tutti noi protagonisti di una discussione intensa e importante, con contributi rilevanti dentro un confronto reale ed articolato che ha portato su alcuni punti a modifiche apprezzabili. Del resto, risultava per noi naturale condividere su questo tema la via del dialogo e del confronto di merito essenzialmente per tre motivi. Innanzi tutto perché quando si parla di riforme delle istituzioni

Un modello che rischiava - questo sì - di accentuare anziché affrontare i profondi divari del Paese perché figlio di una palese confusione. In tutti questi anni al Nord si parlava di federalismo, ma si aveva in testa a volte una vera e propria confederazione di macro Regioni indipendenti e sovrane. Infine, perché c'è una storia tutta nostra su queste tematiche. Il centrosinistra può infatti vantare un'elaborazione lunga, costante e coerente sui temi delle autonomie, della territorialità, del decentramento, dei sistemi locali nel solco dei principi fondamentali e della salvaguardia dei diritti civili e sociali sanciti dalla Costituzione italiana. Siamo tutti consapevoli che la scelta che stiamo compiendo segnerà in maniera decisiva la vita politica, istituzionale, sociale ed economica del nostro Paese. Per questo non possiamo permetterci - non lo potrebbe fare nessuno di noi per la serietà del ruolo che siamo chiamati a svolgere - di ridurre il tutto a propaganda, a demagogia oppure a merce di scambio all'interno della maggioranza per appuntare dei segnaposti sul territorio e per garantire la tenuta di una coalizione intrappolata dai troppo differenti e divergenti interessi che si intendono rappresentare. L'attuazione dell'articolo 119 non può quindi essere un modello ideologico, ma deve rappresentare uno schema di riferimento per progettare una moderna organizzazione dei poteri pubblici, esigenza che dai cittadini viene sentita ed espressa con particolare vigore a causa di una molteplicità di fattori: domanda di maggiore efficienza e trasparenza; controllo dei processi decisionali pubblici; certezza di risorse per gli enti territoriali; individuazione delle responsabilità della spesa; vicinanza al territorio. Esigenze che si coniugano ad un sentimento sempre più diffuso di indisponibilità a vedere che le risorse prodotte finiscano per foraggiare una cattiva amministrazione, di insofferenza verso una dissociazione crescente fra il muoversi dei diritti e il muoversi dei doveri e delle responsabilità, di insostenibilità di un sistema fondato su meccanismi di trasferimenti legati alla spesa storica, fonte di inefficienza, di irresponsabilità e di crescita esponenziale della spesa. E in più, io aggiungo, necessità di rendere esigibili su tutto il territorio nazionale i diritti costituzionali di cittadinanza, oggi palesemente diseguali nel confronto tra territori, al di là del livello istituzionale cui è affidata la competenza. Temi complessi e delicati, che ci presentano la fotografia di un Paese con mali endemici da curare e squilibri forti che hanno radici profonde, per affrontare e superare i quali le classi dirigenti di un Paese dovrebbero essere in grado di spogliarsi delle bandiere e degli *slogan* propagandistici per assumersi, invece, la piena responsabilità di indicare la strada verso il futuro. Ma per prendere una strada e giungere alla destinazione individuata, occorre avere chiaro il punto di partenza, la meta, i mezzi per percorrerla, gli strumenti a disposizione, le caratteristiche del percorso. Con molta franchezza, io credo che, ad oggi, questi punti dirimenti non siano ancora nelle nostre disponibilità. Siamo infatti al paradosso di un federalismo fiscale che il Governo ci presenta senza numeri, senza cifre, senza conti. Stiamo cioè discutendo di una riorganizzazione dei poteri pubblici senza alcuna previsione degli esiti e degli effetti sulla finanza pubblica e sulle singole autonomie territoriali. Mentre si invoca la trasparenza e la certezza delle risorse come uno degli elementi portanti per la costruzione di un rinnovato rapporto Stato-cittadini, ecco che, alla prima prova dei fatti, noi non siamo nella condizione di avere una qualche sorta di simulazione dei dati per comprendere la portata di questo disegno. Siamo altresì al paradosso di una strada che il Governo ha deciso di percorrere in senso inverso: si parte dal punto di arrivo, cioè dalla ripartizione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni e dei servizi

rispetto ai proclami sull'autonomia e sul federalismo che sbandierate sul territorio: l'impianto fortemente centralistico di alcune norme; l'abolizione per il 90 cento del principale cespite di autonomia impositiva locale; il varo in questi giorni di misure in deroga che rappresentano involuzioni gravi e che stanno accentuando il malcontento e moltiplicando confusione e contraddizioni (malcontento che la Lega sta cavalcando con stupefacente disinvoltura nei nostri territori nonostante i suoi rappresentanti a Roma ne abbiano condiviso l'approvazione), e ancora, la debolezza sul tema della lotta all'evasione fiscale, obiettivo che invece dovrebbe essere prioritario considerato che il federalismo fiscale è legato alla ricomposizione della base imponibile, oggi pesantemente erosa dal sommerso e dall'illegalità. In tutto questo, diventa ancor più cogente la modalità con cui affrontiamo la grave e drammatica crisi in atto. Nessuno infatti può pensare che una crisi di queste dimensioni lasci inalterato un quadro politico istituzionale, sociale e culturale. Dalle risposte che diamo, non solo economiche, dipenderà la qualità del futuro del nostro Paese, perché si può uscire da questa crisi o più uniti o più divisi. La crisi determina dei fenomeni che possono minare le stesse caratteristiche di come ci si riconosce nella comunità nazionale e questo rischia di essere tanto più vero in un Paese dove si registrano Prego, E non si tratta solo di disparità tra Nord e Sud, ma anche all'interno degli stessi singoli territori tra chi è più debole e chi è più forte. I segnali in questo periodo non mi paiono certo rassicuranti, se, per esempio, guardiamo alla crescente accentuazione di rivendicazioni corporative e territoriali

trattiene quindi l'83 per cento di quanto paga al fisco. Un impiegato di Mestre versa 12.929 euro all'Agenzia delle entrate e ne riceve indietro 10.147; l'82 A Catanzaro un insegnante versa 6.960 euro e ottiene dallo Stato 10.588 euro, il 151 per cento. La Sicilia riceve il 152 per cento di quanto versa, la Valle d'Aosta il 135 e la Campania si accontenta del solo 126 per cento. Come se non bastassero queste cifre, abbiamo appena concesso 140 milioni di euro a Catania e ben mezzo miliardo di per investimenti, per nuove metropolitane o nuove strade? Assolutamente no, per ripianare i loro debiti. Possiamo puntare il dito contro amministratori locali e responsabili ma temo che troveremmo ampie responsabilità in entrambi gli schieramenti e soprattutto mancheremmo Grazie alla riforma costituzionale del 2001, le Regioni devono farsi carico di un numero consistente di funzioni, senza poter riscuotere tasse ed amministrare il gettito. In sostanza, gli enti locali spendono e poi lo Stato passa a saldare il conto. Non sono solo i cittadini della Sicilia o della Campania a risanare i rispettivi *deficit* sanitari, ma tutti gli italiani e sono stati i soldi dei lombardi, dei piemontesi o dei veneti a tenere accesi i lampioni a Catania e ad evitare il fallimento della capitale. Ebbene, il sistema non funziona, perché, per la quantità di fondi che sono stati distribuiti al Sud, dalla Cassa per il Mezzogiorno ai fondi strutturali europei, la Sicilia dovrebbe essere la *Silicon valley* del Mediterraneo, la Campania il paradiso dei turisti e la Calabria dovrebbe avere un tasso di disoccupazione irrisorio. Così naturalmente non è, e stanziare ulteriori fondi non cambierà la situazione. La Regione Lombardia spende per la sanità 1.695 euro a cittadino, una cifra non molto diversa dai 1.654 euro spesi in Campania o dai 1.639 euro e addirittura meno dei 1.900 euro spesi in Molise. Le cifre sono piuttosto vicine, i risultati che si conseguono con queste somme mi sembrano invece piuttosto distanti.

COLLI *(PdL)*. Le cifre sono piuttosto vicine e i risultati che si conseguono con queste somme mi sembrano invece piuttosto distanti. L'esempio della sanità non è citato a caso: l'83 per cento dei 110 miliardi di euro spesi dalle Regioni ordinarie ogni anno è infatti assorbito dalla spesa sanitaria. Quindi, se non si mette mano a questo specifico settore sarà impossibile qualsiasi contenimento della spesa pubblica. Il disegno di legge sul federalismo che stiamo discutendo in questa Aula tenta di risolvere il problema, stravolgendo il rapporto tra Stato e Regioni. Abbandonando il criterio della spesa storica, lo Stato non avrà più l'onere di rimborsare le Regioni in base a quanto hanno speso fino all'anno scorso, ma garantirà solo il finanziamento integrale di sanità, istruzione e assistenza sulla base dei costi standard, ovvero sulla base di quanto spende per quello stesso servizio una Regione virtuosa. Una TAC costerà la stessa cifra in Molise e in Veneto; un intervento di appendicite non potrà costare in Sicilia quattro volte più di quanto costi in un ospedale piemontese. Se la Regione virtuosa da prendere come riferimento per i costi standard fosse la Lombardia, lo Stato risparmierebbe quattro miliardi e mezzo all'anno (abbastanza per abbassare consistentemente l'IRPEF di tutti gli italiani). L'entrata in vigore del federalismo fiscale comporterà una diminuzione dei servizi offerti nelle Regioni più deboli? Non credo. Credo invece che metterà gli amministratori locali nella condizione di dovere garantire servizi più efficienti senza contrarre debiti infiniti da far pagare al Governo e costringerà i Governatori che vogliono assumere 14.000 forestali a spiegare ai propri cittadini che questa spesa è più utile della costruzione di nuovi asili. Certo, aspettarsi una simile rivoluzione dal testo che stiamo discutendo è forse eccessivo. Il disegno di legge è una delega e i tempi di attuazione saranno naturalmente lunghi. Non si riforma con l'accetta dalla mattina alla sera. L'importante, signor Ministro, è che la riforma non si dilunghi tra riunioni e concertazioni perdendo il suo forte impatto. Già nel 2000 si è tentato di superare il concetto di spesa storica ma, diluendo l'aggiustamento nell'arco di 60 anni, è stato impossibile osservare qualsiasi tipo di beneficio. Spero che la determinazione di questa maggioranza e il momento particolarmente delicato convinceranno molti a ritirare veti e mugugni e a partecipare con orgoglio ad un cambiamento storico del nostro Paese.

Signora Presidente, credo che nessuno in quest'Aula pensi che il nostro Paese, come qualsiasi altra moderna e complessa società contemporanea, possa essere governato come un sistema centralizzato. D'altronde, la formulazione di un ordinamento degli enti locali e del loro finanziamento è un problema aperto in Italia, come in Europa, ormai da decenni. Anche se ciascuno di noi può dare un diverso significato ai principi dell'articolo 119 della nostra Costituzione, che parla di autonomia finanziaria degli enti locali, la questione richiede un grande attenzione. richiede una grande attenzione se ravvisiamo il rischio che la riforma federale possa prendere, nel breve termine, l'indirizzo di una tendenza che somma problemi nuovi a problemi vecchi diventi, come detto più volte in quest'Aula, di difficile comprensione se si è messi nella condizione di parlare, come stiamo facendo oggi, di federalismo fiscale in termini approssimativi nelle grandezze e confuso negli strumenti. strumenti. Prima di tutto, invece, per noi il problema è di un'esatta qualificazione delle competenze, delle prerogative, dei poteri, di previsione di spese autonome e del loro imprescindibile coordinamento con quelle dello Stato: in una parola, paletti rigidi per tenere insieme solidarietà e responsabilità. Senza pregiudiziali ideologiche o tecniche (per questo motivo questa mattina non abbiamo posto la questione pregiudiziale), ma solo con una volontà positiva e e propositiva, riteniamo sia fondamentale prima di fare delle scelte - come ricordato anche dal relatore dell'opposizione - disporre di una base di dati condivisi sulle entrate, sulle uscite, sui flussi, sul debito e sulle dinamiche aggregate:

Certo, il testo è stato molto cambiato dall'inizio della discussione presso le Commissioni riunite. Si è passati da un federalismo «ognuno per sé», modello lombardo, ad un disegno di legge che almeno nelle intenzioni dovrà garantire la copertura dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali sul territorio, anche se molti di noi sanno che fine hanno fatto i livelli essenziali nel settore della sanità. Ma poiché nonostante tutto per il momento è presente solo uno schema di princìpi, mancando i numeri che solo i decreti delegati di attuazione potranno riempire, resta per il Paese un problema di fondo rappresentato dalle risorse economiche, dai soldi. Bisognerà capire quali cifre corrispondonoai princìpi enunciati, verificare punto per punto le risorse e i servizi per i cittadini in tutto il Paese. E in questo senso la crisi economica e la recessione che attraversa il Paese non aiuta affatto, anzi complica e rende sempre più fragile la solidarietà tra i territori, tra Nord e Sud, e non crea certo un ambiente favorevole all'attuazione del federalismo, perché ci saranno meno risorse per attenuare e attutire il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

ora, con la crisi economica internazionale, a chiedere più autonomia fiscale sono rimaste solo le regioni più ricche. Malgrado, quindi, la complessità di questo quadro, di cui ci rendiamo conto, vorremmo che fossero chiari almeno la riforma nella sua interezza deve essere condivisa dal Parlamento. Il nodo centrale da risolvere è proprio questo da altri che mi hanno preceduto: un adeguato coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione dei decreti delegati di attuazione, contemperando il ruolo del Parlamento con quello delle autonomie.

parlamentari, non potrà certo assicurare un giusto equilibrio. Un secondo punto fermo è che l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe andare di pari passo con quella del federalismo istituzionale, non per rinviare il problema

Untema importante, che è stato ricordato, appare la trasformazione del Senato in una vera e propria Camera delle Regioni deputata ad un ruolo di raccordo tra i diversi livelli di Governo nel nuovo sistema federale. federale. Altrettanto importante sarà poi alleggerire la lunga gerarchia di enti di governo territoriale, abolendo - come si era tutti d'accordo in campagna elettorale - le Province. è importante che si faccia chiarezza su chi fa cosa tra i vari livelli di governo e che non sia mantenuta estesa l'area delle competenze concorrenti tra più livelli: infatti, è evidente che quanti più livelli di governo hanno competenza su una stessa materia, tanto più diventa difficile tenere ferme le precise responsabilità di ciascuno. Un terzo punto chiaro e fermo è che bisogna evitare un federalismo alla rovescia, con una logica invertita.

Partendo dalle entrate si rischia non solo di incoraggiare l'aumento della spesa pubblica, soprattutto in quelle Regioni la cui capacità fiscale eccede il fabbisogno delle spese, ma anche di compromettere la stabilità delle finanze statali. Il bilancio dello Stato resta in disavanzo e non vi sono risorse libere da trasferire. Il federalismo non può indebolire la responsabilità collettiva per il servizio del debito pubblico e per la copertura delle spese per i servizi statali (come il sistema previdenziale). Cari colleghi, noi rischiamo di produrre un federalismo fantasma se non si chiarisce da subito e non si precisa cosa si intende per fabbisogno standard, individuando gli indicatori tesi a definire la necessità in termini di servizio per una data Regione (e quindi dei relativi riferimenti), che non possono essere solo dei parametri demografici o di rapporto tra dipendenti pubblici e residenti, parametri di delicata valutazione, come quelli socio-economici. Nel nostro Paese è evidente una forte variabilità territoriale nella spesa per i servizi sociali, particolarmente accentuata nel caso di servizi delicati, legati all'assistenza, alla beneficenza, agli asili nido. Un esempio significativo: la spesa *pro capite* per i servizi sociali in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata è del 50 per cento inferiore a quella della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, della Liguria, dell'Emilia-Romagna, della Toscana. Ciò che colpisce è il disallineamento rispetto alla domanda potenziale collegata ai fattori demografici: cioè, le differenze territoriali sono spesso di segno opposto rispetto alla domanda attesa, perché tale domanda è legata ad indicatori di disagio economico, quali il tasso di povertà o quello di disoccupazione, o è legata altre volte, per i servizi all'infanzia, al minor tasso di occupazione femminile nelle Regioni meridionali, e altre volte ancora, per l'erogazione dei servizi a favore degli anziani, al maggior ruolo che nelle Regioni meridionali la famiglia riveste nell'ambito delle cure agli anziani stessi. Nel disegno di legge in esame non vediamo inoltre, signor Ministro, un impegno preciso di invarianza fiscale. Anzi, il rischio è che, spostando a livello locale l'effetto di progressività dell'imposta, possano crearsi distorsioni sul territorio nazionale e incentivi a spostamenti verso realtà a più basso prelievo: una sorta di esodo fiscale. C'è quindi il pericolo di un aumento della complessità e della scarsa trasparenza del sistema fiscale: il cosiddetto fenomeno della regionalizzazione dell'IRPEF. Un altro aspetto problematico è rappresentato dall'attuale assetto del Patto di stabilità interno, che per le Regioni ha come aggregato di riferimento non più un saldo di bilancio, ma un aggregato di spesa. Così come gli obiettivi Così come gli obiettivi di bilancio fissati per gli enti locali fanno riferimento ad un saldo che include gli investimenti e quindi, per loro natura, non sono comprimibili senza alterare lo stesso equilibrio di bilancio. Insomma, il federalismo fiscale non è la panacea di tutti i mali, a maggior ragione nel campo dell'occupazione. Il federalismo da solo non potrà bastare a colmare il divario occupazionale tra il Nord e il Sud. Per questo, a nostro giudizio, occorrerà introdurre al Sud misure come la fiscalità di vantaggio e la possibilità di differenziare il costo del lavoro. Collega, la prego è una confusa sommatoria di rivendicazioni, in cui ognuno accampa per sé pezzi di risorse più o meno riferite al proprio territorio, perdendo di vista quel disegno riformatore che serve ad unire il Paese: ad unirlo però, signor Ministro, in una maniera diversa rispetto al passato.

rinviabile e vitale, se non vogliamo assistere all'inevitabile e definitivo collasso dei suoi assetti istituzionali.

con uno scarto di soli quattro voti dal Governo delle sinistre nel 2001 senza, peraltro, preoccuparsi di dare attuazione concreta all'articolo 119 della Costituzione. È questo l'asse mancante dal quale sono in larga misura poi dipesi la farragine di competenze, la deresponsabilizzazione amministrativa ed i paralizzanti conflitti tra i vari livelli istituzionali che sono seguiti da quella legge e che il Paese ha pagato e sta continuando a pagare a caro prezzo. E non v'è chi non sappia che si tratta di una situazione alla quale bisogna porre subito un apposito rimedio, come da tempo peraltro la stessa Consulta ha evidenziato con numerosi richiami. Ma è di oggi una notizia che trovo particolarmente interessante per il dibattito generale su questo provvedimento di così rilevante portata. Ed è l'esito di un sondaggio fatto dalla Confcommercio-Format secondo il quale il 62,4 per cento degli italiani ritiene il federalismo una riforma che serve veramente al Paese. Anzi, secondo la ricerca, il 66,2 per cento si dichiara favorevole al decentramento delle strutture dello Stato, per cento ritiene che le Regioni più deboli debbano essere aiutate da quelle più forti e l'87,3 per cento giudica positivamente la possibilità degli enti locali di gestire autonomamente le risorse del proprio territorio. per cento poi, ci dicono le indagini svolte da questa statistica, il federalismo è un possibile veicolo di rinnovamento della democrazia nel nostro Paese, cento prevede che porterà ad una pressione fiscale inferiore o, al peggio, uguale a quella attuale e il 58,7 per cento prevede, addirittura, un miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati. Che il federalismo fiscale sia necessario e, al contempo, anche un'occasione storica per riformare in profondità e in meglio gli assetti del Paese per modernizzarlo e per creare finalmente ad ogni livello istituzionale condizioni di amministrazione della cosa pubblica trasparenti, responsabili e pienamente comprensibili e palpabili, valutabili da ogni cittadino è, dunque, ormai largamente convinta anche l'opinione pubblica nazionale. E questo è un primo fatto. Il secondo è che la qualità dell'impianto e dei contenuti del disegno di legge delega, comprovata dalla convergenza e dal sostanziale apprezzamento già espresso da tutti i livelli di governo interessati (Conferenza Stato-Regioni, ANCI) e scaturita da quel percorso di confronto - che ha voluto riconoscere nel suo intervento in Aula stamattina anche il relatore di minoranza, senatore Vitali - che ha registrato un'apertura corretta e leale nella maggioranza alle valutazioni dell'opposizione, evidenzia tra l'altro anche il lavoro faticosissimo delle tre Commissioni parlamentari animate da un lavoro appassionato, equilibrato, guidato dalla riconosciuta competenza del presidente Azzollini e dei presidenti Vizzini e Baldassarri. con pazienza certosina e vincendo molte resistenze, spesso pregiudiziali, il ministro Calderoli, da una parte, e il ministro Fitto, dall'altra (quest'ultimo soprattutto con un intenso, quanto delicato e discreto lavoro di tessitura e di confronto istituzionale con le Regioni), hanno condotto un'opera eccellente producendo un testo che può davvero rappresentare il punto di svolta per cambiare il Paese, combattere le inefficienze, responsabilizzare gli amministratori e i cittadini e dare quello slancio necessario per rilanciare lo sviluppo dell'economia e restituire ai cittadini fiducia per il futuro e anche rispetto per la politica e per le istituzioni. Trovo solida l'architettura complessiva del provvedimento, così come anche è stata migliorata attraverso la fase emendativa nelle Commissioni di merito. Ciò permetterà che l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria - fra le altre cose - da parte delle Regioni, ovviamente nelle materie non assoggettate alla competenza dello Stato, determini effetti di ricaduta assolutamente positivi, caratterizzati da una fase transitoria e progressiva, capace di restituire razionalità alla distribuzione delle risorse e di renderle coerenti con il costo standard delle prestazioni erogate. In questo senso è decisivo il superamento del criterio della cosiddetta spesa storica, che tanti disturbi sta producendo soprattutto in alcune Regioni che, dai criteri del provvedimento Bindi, per quanto attiene alla suddivisione del fondo, hanno in effetti ottenuto una riduzione in ordine ai relativi e rispettivi bisogni. Si tratta di un aspetto che, sostituito con parametri di spesa standard, sulla base di obiettivi che tengano conto dei relativi costi di soddisfacimento, in un confronto equilibrato e perequato attraverso l'apposito fondo previsto all'articolo 7 (sancito peraltro attraverso princìpi verticali), consentirà il rilancio su tre punti fondamentali nel percorso delle politiche sociali e di *welfare*: mi riferisco in particolare alla salute, all'istruzione e ai servizi sociali. per quanto riguarda il principio della territorialità nell'attribuzione dei gettiti, si tratta di una leva fondamentale per sensibilizzare e al contempo responsabilizzare le amministrazioni locali. In proposito - e lo dico da parlamentare del Sud debba essere proprio il Sud a cogliere questa come una vera opportunità, che può essere tale e può aprire una svolta nel miglioramento dell'efficienza del territorio del Mezzogiorno, nel momento in cui si saprà realmente ricongiungere l'onore della spesa con l'onere della tassazione. Un secondo aspetto riguarda il metodo che è stato seguito: ci sono tre importanti articoli (il 3, il 4 e il 5) che prevedono la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che consentirà l'approfondimento

permanente per il coordinamento della finanza pubblica, aspetto questo particolarmente rilevante, perché tutela il rispetto di due principi costituzionalmente sanciti: quello dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini riguardo ai servizi rilevanti per il godimento dei diritti civili e quello della buona amministrazione. Ha ragione, infatti, il collega senatore Astore: questo non può che essere considerato un percorso normativo che pone fine agli egoismi localistici e nel quale non sono penalizzati gli amministrati, ma gli amministratori che sbagliano. Concludo, signora Presidente, dicendo che i princìpi di equità, di efficienza e di logica solidale, uniti al necessario recupero di una politica sociale omogenea sul territorio nazionale, in cui non c'è più chi è forte e chi è debole, ma c'è un principio di assoluta equità, passano dalla strada stretta e difficile della responsabilità, che non può e non deve più tollerare che le risorse economiche pubbliche servano a finanziare le inefficienze o, peggio, ad utilizzare il potere politico, amministrativo e gestionale che riesce a deviare illecitamente le risorse finanziarie per disinvolti sistemi di clientela elettorale. Con prudenza ed equilibrio, signora Presidente, ma anche con grande determinazione, diciamo che la ricreazione è finita: è una svolta negli assetti istituzionali del Paese, ma è anche una vera e propria sfida culturale per l'intero Paese.

Da un punto di vista politico, va riconosciuto che il testo al nostro esame, sin dal principio, si è presentato molto aperto ai diversi contributi di Regioni, enti locali, parti sociali (su ammissione stessa del ministro Calderoli), al punto tale che taluni ritengono ne sia risultato un testo in molti punti addirittura contraddittorio.

dovrebbe ormai essere chiaro a tutti: si tratta del passaggio dal criterio della spesa effettiva a quella standard ovvero dell'obiettivo di sostituire gradualmente, a tutti i livelli (Regioni ed enti locali), il sistema di finanziamento di alcune funzioni pubbliche basato sulla spesa effettiva con la spesa standard. Rispetto al testo iniziale proposto dal Governo, vanno poi segnalati (senza elencarli in quanto già precisamente descritti nella relazione di accompagnamento al testo approvato dalle Commissioni) gli elementi di novità apportati in Commissione: dall'indicazione di un riferimento preciso per l'autonomia tributaria degli enti locali all'armonizzazione dei bilanci pubblici, all'introduzione del metodo della programmazione pluriennale per gli interventi speciali per la coesione e il Mezzogiorno. restano tanti punti inevasi, a cominciare, per il Mezzogiorno, dalla fiscalità di sviluppo, inserita tra i criteri direttivi dell'articolo 2, che però probabilmente non potrà essere di particolare ausilio per le Regioni più deboli, in quanto la giurisprudenza comunitaria ha recentemente chiarito che le entità sub-statuali devono, in pratica, autofinanziarsi la fiscalità di sviluppo. soprattutto inevaso il problema politico di fondo relativo all'impostazione che si vuole dare a questo disegno di riforma per far sì che sia ben accetto dagli italiani, come la maggioranza (della quale io faccio parte) si augura, volendo esprimere una condivisione consapevole del testo e non conferire un mandato acritico, un sì strappato, *obtorto collo*. Non credo che il federalismo fiscale possa essere qualcosa di diverso da un gioco a somma zero ovvero un gioco in cui alcuni soggetti istituzionali perdono qualcosa ed altri guadagnano. Nello schema proposto, auspicabilmente tra i primi vi è lo Stato centrale e la parte di spesa pubblica che viene ridotta è quella che adesso viene dilapidata in spese inutili, improduttive e clientelari. Così invece purtroppo non è; sembra quasi che tutti ci guadagnino in questo processo. A leggere le cronache degli ultimi mesi, si registrano le dichiarazioni dei Presidenti delle Regioni speciali, in particolare del Trentino, della Sicilia e della Sardegna, quelle dei sindaci del cosiddetto club del 20 per cento dell'IRPEF, quelle dei sostenitori di Roma capitale, quelle dei Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno (segnatamente, la Calabria e la mia Campania) e quelle dei Comuni confinanti con le Regioni speciali. In altre parole, così procedendo, il federalismo contrattato rischia di essere snaturato *in nuce*, per essere affidato, anche nella fase attuativa, ai mutevoli orientamenti dei responsabili dell'attuazione del processo, innescando un processo emulativo tra territori, che è l'esatto contrario del processo virtuoso che invece dovrebbe portare a ridurre la spesa improduttiva e quindi, di conseguenza, la pressione fiscale. Un esempio è dato dall'attuazione che si intende dare alla previsione degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della nostra Costituzione. Non so, infatti, se il riferimento, contenuto nell'articolo, ai territori di confine o confinanti con Regioni di confine destinatari degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto, della Costituzione, sia veramente rispettoso dello spirito della Carta costituzionale, che evidentemente è rivolta a territori svantaggiati e ad esigenze speciali di perequazione infrastrutturale. Ora, non vi è dubbio che in Italia occorra maggiore autonomia fiscale da parte degli enti locali e delle Regioni, ma vi è da temere da una interpretazione di tale linea in chiave di «federalismo esploso e competitivo», dove in pratica ciascun livello di Governo si sente legittimato ad autogovernarsi in termini finanziari pretendendo, *ex post*, il ripiano finanziario al di fuori di una logica nazionale. A riprova di ciò sta proprio l'«andazzo» - per così dire - certamente non commendevole di questi anni, con ripiani a piè di lista e concessioni *una tantum* a singoli enti. Ciò genera, già oggi, sprechi, sovrapposizioni, costose competizioni in luogo di virtuose cooperazioni, moltiplicazione di iniziative e di normative, dissesti finanziari e imprese temerarie, come l'uso spregiudicato, se non colpevole, dei prodotti finanziari derivati. Io che vivo in Campania e seguo le vicende della mia Regione ne ho - ahimè - conoscenza. In questo quadro, certamente il superamento del criterio della spesa storica dei trasferimenti attraverso la definizione dei costi standard dei servizi essenziali, in modo da premiare i comportamenti virtuosi e limitare gli sprechi e la cattiva amministrazione, è un principio commendevole; ma si tratta di qualcosa che era già sperimentato all'estero, prima che in Italia nella sanità. In pratica, è però poco più che un modello, certo positivo, ma di programmazione pubblica. Molto più opinabile è il passaggio successivo che affida alle Regioni le decisioni in ordine al loro contributo alla perequazione. Mi riferisco, ovviamente, al fatto che la definizione dei costi standard che dovrebbero guidare la perequazione territoriale delle risorse rinvia il problema politico fondamentale della distribuzione delle risorse sul territorio nazionale alle decisioni

Non posso non chiedermi, a questo punto, sperando di essere contraddetto dai fatti, quale possa essere l'esito, in questo contesto, del processo di federalismo per le Regioni più deboli del Sud. A rischio di apparire pedante, signora Presidente, non posso non ricordare alcuni dati economici del nostro Sud. Il tasso di occupazione della popolazione tra i 15 e i 64 anni è del 65-70 per cento nel Centro-Nord, mentre è del 42-50 per Due terzi delle famiglie povere sono al Sud. Il reddito *pro capite* del Sud è circa il 75 per cento di quello del Centro-Nord, e quello della Regione più ricca (la Lombardia) è circa due volte quello della più povera (la Calabria). A fronte di ciò, per le entrate si registra invece una distribuzione territoriale della spesa abbastanza uniforme sul territorio nazionale: da qui il prodursi dei predetti residui fiscali. Per questo motivo ho inteso avanzare una proposta emendativa che si prefigge lo scopo di provvedere al bilanciamento del criterio della territorialità per la compartecipazione da parte delle Regioni ai tributi erariali (essenzialmente, l'IVA), che trovano la loro base imponibile sui consumi, con il vincolo di determinazione della misura dell'aliquota della compartecipazione con l'effettiva capacità fiscale delle Regioni, considerate le caratteristiche delle basi imponibili e fondandone la misura in relazione ad un paniere di beni che sia il più possibile omogeneo su tutto il territorio nazionale. Non vi è chi non veda, infatti, come l'applicazione acritica ed esclusiva del solo criterio della territorialità alla compartecipazione delle Regioni ai tributi erariali su tutti i consumi, indipendentemente da un ambito applicativo che tenga in debito conto la qualità dei beni e servizi su cui incidono gli stessi tributi, potrebbe comportare il perverso effetto di avvantaggiare oltre misura le Regioni per cui, dati i livelli di reddito sensibilmente superiori alla media nazionale, il livello dei consumi voluttuari e, in genere, di beni e servizi superiori rispetto a quelli primari...

anzitutto sul terreno civile e delle virtù morali delle comunità, ed è su ciò che qualsiasi politica di sviluppo deve, prima di ogni altra cosa, puntare. In ciò, e non nel mero assistenzialismo, si concreta quel principio di solidarismo che deve guidare le politiche di sviluppo del Mezzogiorno. Come, infatti, ebbe a dire Alcide De Gasperi (presidente del partito dal quale provengo, la gloriosa Democrazia cristiana) nel 1953: «Il solidarismo è quel sistema sociale che eleva a principio della convivenza umana la solidarietà di ogni comunità con i suoi membri, e dei suoi membri con la comunità». Non si tratta di essere sordi alle istanze di quanti intendono introdurre criteri di controllo del finanziamento alle funzioni pubbliche più attenti alle esigenze di efficienza

Signora Presidente, colleghi, intervengo con lo spirito di chi vuol dare un contributo essendo appassionato del tema del federalismo fiscale per la Regione da cui provengo, la Lombardia.

quindi, con lo spirito di chi attende da tempo di vedere in Parlamento approvata una legge sul federalismo fiscale. Stiamo parlando di federalismo fiscale, non già di Stato federale: questo è importante dirlo.

Dobbiamo camminare con questo provvedimento con i piedi per terra, non creare eccessive illusioni. Sappiamo come in Lombardia e in tutto il Nord ci sia molta attesa per questo provvedimento e come questa non vada delusa neanche creando castelli per aria. aria. Non evocherei neanche, quindi, grandi modifiche costituzionali; camminerei proprio diritto verso l'obiettivo: cerchiamo di realizzare nel più breve tempo possibile l'approvazione di questa legge essendo frutto, tra l'altro, di una collaborazione utile e positiva dentro il Parlamento; cerchiamo di farlo in modo condiviso anche nella Commissione che dovrà valutare i decreti delegati. È chiaro che ammodernare la pubblica amministrazione - lo abbiamo detto tutti oggi nel proficuo dibattito che c'è stato tra centrodestra e centrosinistra - significa rendere più efficiente ed efficace la spesa pubblica; significa rendere comprensibile la relazione fra le tasse pagate e i servizi erogati in termini di qualità e quantità; significa identificare il più possibile il luogo dell'imposizione fiscale con quello della spesa pubblica, avvicinando il più possibile questo È stato detto da tutti, tra l'altro, che bisogna realizzare ciò recuperando il senso della responsabilità dell'amministrazione pubblica rispetto al denaro speso. Si tratta di ridurre gli sprechi, migliorare la qualità dei servizi e, quindi, rendere di fatto più eguale il nostro Paese. Oggi non è così; sappiamo che ci sono profonde differenze anche laddove - penso alla sanità - una progressiva regionalizzazione dei servizi è stata approvata. Vi

Sono più appassionato dell'autonomia locale che non del regionalismo; penso che non dobbiamo fare grandi modifiche costituzionali, ma una revisione del Titolo V per quanto riguarda le materie concorrenti forse dovremmo avvicinarci a farla, perché questa conflittualità fra Stato e Regioni spesso crea situazione di stallo. Si tratta di stabilire livelli standard dei servizi essenziali e il costo di questi servizi, superando la concezione di costo storico e facendo, quindi, un passo avanti fondamentale. fondamentale. Questi principi in questo disegno di legge delega ci sono ed il suo contenuto è anche frutto di un lavoro condiviso. Penso che il Partito Democratico abbia dato un utile contributo; speriamo di poterlo dare ancora. abbiamo contribuito anche all'idea solidale del meccanismo federale che stiamo mettendo in piedi. Idea solidale significa attivare meccanismi perequativi che superino, quindi, quel concetto un po' egoistico contenuto nella legge proposta dal Consiglio regionale della Regione Lombardia e, in un primo momento, anche dalla Lega Nord. Sicuramente tutti insieme abbiamo fatto un percorso

Certo che, se questo provvedimento è condivisibile nel suo impianto fondamentale, il rischio è che, oggi come oggi, rimanga però un esercizio accademico o perlomeno un esercizio legislativo fra di noi, perché bisogna capire anche cosa c'è dietro questi princìpi comunemente espressi, cosa c'è sotto il vestito che abbiamo confezionato. Questo ancora non si capisce bene, il Governo non è riuscito a spiegarcelo, perché capire se l'ammodernamento che stiamo disegnando diventerà realtà o un pasticcio è un discrimine importante: oggi non si riesce ancora a comprenderlo, dipenderà dai decreti delegati e da come lavoreremo in futuro. Quale sarà il risultato economico che le autonomie locali porteranno a casa ancora non è chiaro. Oggi una cosa è chiara: che l'ICI non c'è più, che i trasferimenti che dovevano sostituire l'ICI non sono sufficienti,

D'altra parte, nei fatti, con un Governo che sta togliendo risorse agli enti locali c'è questa contraddizione, che in qualche modo va risolta se vogliamo essere credibili fino in fondo, altrimenti resta un libro dei sogni, non realizzabile; mancano le risorse per realizzare quello che c'è scritto. Il Governo questo ancora non ce lo ha detto. Teniamo presente che facciamo questo disegno di legge non per creare venti Stati in più ma per dare più forza alle autonomie locali; facciamo un federalismo fiscale, non un federalismo regionale. Questo è importante dirlo e riaffermarlo.

alcune cose buone e alcune ombre, che spero che il Governo riesca a fugare, soprattutto nel percorso che dobbiamo ancora fare insieme valutando i decreti delegati nelle Commissioni che li esamineranno. possa proseguire e che il federalismo non sia solo una bandierina sventolata sul pennone della propaganda politica, ma che possa diventare una realtà proficua e utile allo sviluppo del nostro Paese. Signora Presidente, signori colleghi, signor rappresentante del Governo, non so se oggi sarà una giornata storica, com'è

Devo innanzitutto dare atto al relatore Azzollini, al ministro Calderoli, al ministro Bossi e al sottosegretario Brancher di aver fatto un prezioso lavoro di sintesi e di mediazione. Sono molto meravigliato che il ministro Calderoli sia arrivato, dopo i tempi delle sue rigidità, a svolgere un ruolo di grande mediatore, ma questo testimonia il fatto che i tempi cambiano profondamente. Credo che le mediazioni trovate sul provvedimento in esame consentano oggi a tutte le forze politiche di centrodestra e alle forze politiche anche dell'opposizione di esprimere un giudizio tendenzialmente positivo, anche se sarà un giudizio di astensione. il disegno di legge, sul piano anche di una certa ambiguità, un provvedimento che oggi consente a tutti di riconoscersi; un provvedimento che consente a coloro che vengono dal Nord e che lo hanno sostenuto (*in primis* la Lega, ma le Regioni del Nord in particolare, che si sono battute sulla questione del federalismo fiscale) di riconoscersi e di sperare che attraverso lo stesso finalmente una parte considerevole del gettito fiscale proveniente da queste aree, che sono le aree più produttive e dinamiche del nostro Paese,

sia pure di fronte a delle modifiche che verranno introdotte, si giocherà una partita ancora valida sulla redistribuzione della fiscalità del nostro Paese.

emergeranno successivamente quando si andranno a definire i decreti delegati. A quel punto si capirà veramente che tipo di partita si giocherà.

La definizione dei cosiddetti costi standard e del conseguente fabbisogno finanziario è una questione che sul piano teorico è facile da risolvere, ma sul piano pratico è davvero complessa. Non si può pensare che i costi standard siano omogenei su tutto il territorio nazionale: i costi per fornire certi servizi sono differenziati, diversificati a seconda che si operi al Centro, al Sud o al Nord e di questo si dovrà tenere conto. Ma il secondo problema fondamentale, sul quale credo si innescherà un confronto territoriale molto consistente, è quello della costituzione e dell'alimentazione finanziaria del fondo perequativo,

o Emilia Romagna, nonché della spesa complessiva - che deriva sia dalle amministrazioni centrali dello Stato, cui faccio rientrare anche gli enti pensionistici, dal debito pubblico e dal sistema aggregato delle amministrazioni locali

Contestualmente è accaduto un fenomeno di cui occorre tener conto. In questi anni le Regioni che hanno avuto la fiscalità maggiore e sono stati i massimi gestori della solidarietà nazionale hanno

che gestisce maggiormente questa politica di solidarietà, ha avuto una riduzione del PIL, tra il 2000 e il 2005, del 6,3 per cento; la Lombardia del 2,7 per cento e il Veneto dell'1,9 Tutto sarebbe giustificabile, in una politica di riequilibrio e di ridefinizione dei rapporti Nord-Sud, se contestualmente, per i notevoli trasferimenti realizzati nel Sud, il prodotto interno lordo *pro capite* delle Regioni La verità è che purtroppo in larga parte delle Regioni del Sud non è cresciuto, salvo la Sardegna e il fanalino di coda (ma è molto relativo) che è la Calabria; per il resto, il prodotto interno lordo *pro capite* è sceso anche in queste aree. Quindi, con questa redistribuzione della fiscalità del nostro Paese, non abbiamo avuto una politica di sviluppo delle aree svantaggiate rispetto a quelle ricche. ricche. Il problema che mi pongo, e su questo si scateneranno tutte le contraddizioni, è il seguente: le regioni ricche del Nord - soprattutto in una fase storica come quella attuale di forte crisi economica, di riduzione del del prodotto interno lordo, di anni difficili come quelli che si appalesano di fronte a noi - con i meccanismi che abbiamo introdotto per la costituzione del fondo di perequazione, continueranno ad alimentarlo come partecipazione al gettito dell'IVA o dell'IRPEF?

e la prima a Statuto ordinario, dove il sistema di trasferimenti di funzioni, di trasformazione e compartecipazione al gettito dei maggiori tributi è già stato realizzato.

comincerà a ragionare pesantemente sull'opportunità di mettere a disposizione risorse per il riequilibrio territoriale. Su questo scatteranno tante contraddizioni e la mia preoccupazione è che

la possibilità di riequilibrio o di mediazione tra gli interessi contrastanti del Paese possa venire meno. Infine, due ultime considerazioni: non

l'autonomia speciale dico che ciò non è vero. Però, mi pongo la questione che le stesse Regioni a Statuto speciale debbano concorrere per la loro quota-parte a costruire un sistema più efficiente, in quanto anche nelle Regioni a Statuto speciale ci sono inefficienze, sprechi, disuguaglianze di gestione che vanno modificate. Se la ristrutturazione del Paese deve essere complessiva devono partecipare anche le Regioni a Statuto speciale.

*(PdL)*. Illustri, resistenti e pazienti senatori, il noto filosofo libanese Gibran Khalil Gibran diceva che l'ovvio è quello che non si vede mai finché qualcuno non lo esprime con la massima semplicità. Nel caso del nostro Paese l'ovvio è la netta differenza sul piano dello sviluppo che esiste tra i diversi territori che lo compongono. Può realizzarsi lo sviluppo armonico di un Paese se il suo territorio è cresciuto in maniera disarmonica? È possibile parlare di prestazioni e di costi standard dello Stato se le sue infrastrutture non si sono sviluppate armonicamente, o se la capacità reddituale o fiscale di ciascun cittadino non è standardizzata né al momento standardizzabile? È possibile standardizzare l'apporto di un territorio allo sviluppo di uno Stato se tra i territori che lo compongono esistono livelli di occupazione, di disoccupazione molto diversi tra loro così come molto diversi tra loro sono i tassi di infrastrutturazione? Le risposte a queste domande apparentemente retoriche sono scontate. La standardizzazione di un risultato in termini di prestazioni o costi non costituisce affatto una variabile indipendente dalla standardizzazione di tutti quei fattori che interagiscono con il risultato che si intende ottenere, risultato che non è affatto sganciato dalla storia di quel Paese e dei suoi territori,

alla luce di circa centocinquant'anni anni di politiche unitarie e di oltre sessant'anni di democrazia repubblicana, un periodo quello descritto, nel corso del quale il volto dell'Italia è molto cambiato, anzi si è proprio capovolto a vantaggio di alcuni ed a svantaggio di altri. Il collega Izzo ha citato i dati socio-economici attuali, io vi parlerò brevemente di quelli risalenti agli anni precedenti l'Unità d'Italia.

Pensate, che su 180 milioni di alberi di ulivo, signor relatore, 50 milioni erano nella sua Puglia e che gli opifìci del settore agroalimentare erano oltre 1000. Pensate che il 55 per cento della forza lavoro in agricoltura ed il 51 per cento della forza lavoro nell'industria era al Sud e che al momento dell'Unità d'Italia la riserva aurea del Paese ammontava a 671 milioni di lire dell'epoca, di cui 444, pari a due terzi, al Sud. Pensate che al Sud aveva sede la più grande industria metalmeccanica, il più grande cantiere navale, la più grande industria siderurgica, i più grandi allevamenti di bestiame, la più grande cartiera, la più importante casa editrice e la prima ferrovia. Al Sud fu impiantata la prima illuminazione a gas ed istituito il primo corpo dei vigili del fuoco. Persino il primo codice marittimo fu redatto al Sud. onorevoli colleghi, è più lunga di quella che si racconta, soprattutto più lunga di quella che ho sentito in quest'Aula in queste ore. Se, a distanza di circa centocinquant'anni anni la situazione, invece che bilanciarsi, si è invertita, vuol dire che qualcosa non ha funzionato; vuol dire dunque che qualcosa deve essere corretto o forse che qualcuno ha rubato. Oggi il Sud si trova in una condizione di arretratezza del tutto insopportabile e questo se è, in parte, effetto di una classe dirigente inidonea e prona, per altro verso non può che essere l'effetto di macroscopici errori compiuti nelle politiche pubbliche praticate dallo Stato centrale e dai partiti centralistici. Oggi, parlare di federalismo fiscale significa riallineare ed armonizzare la situazione economica, sociale ed occupazionale di tutti i territori italiani, compiendo uno sforzo, in termini di regole, comportamenti e coraggio, per nulla indifferente, ma facendo chiarezza su quella che è stata la storia di questo Paese. Lo Stato, è vero, costa troppo e produce poco; gli sprechi sono tanti e del tutto immotivati; la qualità della vita è diversa e sperequata. Il federalismo fiscale di cui parliamo, dunque, non costituisce soltanto la concreta attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, come ha più volte chiesto la Corte costituzionale, ma anche lo strumento attraverso il quale ridimensionare i costi dello Stato ed il peso fiscale sui cittadini e le imprese e responsabilizzare i livelli di governo dei vari territori, sia sul piano regionale sia sul piano provinciale e comunale. Infatti, perpetrare un modello di sostanziale finanza derivata in un Paese che con la riforma costituzionale del 2001 ha decentrato numerose competenze legislative crea problematiche di notevole rilevanza (come ben sappiamo noi siciliani per statuto abbiamo competenze diverse dalle altre Regioni, senza avere spesso ottenuto i relativi compensi perequativi per quelle

situazione istituzionale che produce a sua volta l'ingovernabilità dei conti pubblici, la duplicazione delle strutture, l'inefficienza e la deresponsabilizzazione, effetto quest'ultimo che confonde anche il giudizio sull'azione politica e amministrativa che i cittadini hanno il diritto‑dovere di esprimere con il loro voto. Ripianare a piè di lista i conti delle amministrazioni inefficienti, come accaduto con il criterio della spesa storica, è del tutto incompatibile con i principi della sana amministrazione, così come è profondamente ingiusto che chi ha più speso possa continuare a farlo a scapito di chi ha meno e meglio speso. Onorevoli colleghi, il Governo, le Commissioni 1a, 5a e 6a e il relatore legge, il senatore Azzolini, operando in sinergia tra maggioranza e opposizione e in armonia con le risorse disponibili e con gli altri attori del processo federalistico, hanno dato vita ad un testo assai equilibrato che costituisce la cornice all'interno della quale si muove la delega che conferiremo al Governo stesso in materia di federalismo fiscale. Si tratta, come dicevamo, di un provvedimento coraggioso assunto nell'ottica di un'attenta armonizzazione della qualità della vita, dei costi, dei fabbisogni, dei servizi e delle infrastrutture in tutti territori del Paese, nella consapevolezza che è necessario e urgente superare tutti gli errori del passato. Mi riferisco soprattutto a quelli che hanno provocato purtroppo quell'assurda e colpevole inversione di tendenza nei processi di sviluppo del Nord e del Sud da 150 anni a questa parte e di cui ho già detto. Mi riferisco ai meccanismi perequativi, che non possono giammai essere considerati sostitutivi di quelli ordinari (come accadde con la truffa negli anni Sessanta

perequazione medesima e mi riferisco al rispetto delle prerogative statutarie delle Regioni autonome, come prevede il testo elaborato dalle Commissioni congiunte sulla base di un apposito emendamento accolto dal Governo. signor Ministro, onorevole Presidente del Senato, è sulla reale capacità perequativa che si gioca la partita dello sviluppo armonico del Paese, ma all'interno del concetto stesso di perequazione assume un valore assoluto la perequazione infrastrutturale, su cui personalmente ho molto lavorato insieme ad alcuni colleghi, pazienti come me, e presenti qui stasera, quali il senatore Alicata e il presidente Azzollini. Se in uno Stato gli indici quantitativi, per unità di territorio o di abitanti, riguardanti le ferrovie, le strade, le autostrade, le reti elettriche, le reti di distribuzione del gas, le reti fognarie, il numero di aule scolastiche non sono allineati tra loro, non è ipotizzabile pensare a nessuna standardizzazione, né di costi, né di fabbisogni. È per questa ragione che, insieme ad altri colleghi, mi sono soffermato sul tema, con un emendamento interamente accolto dal Governo (l'articolo 21 del testo), per il quale ringrazio il ministro Calderoli. da uomo del Sud, ringrazierò di più l'intero Governo se opererà in modo tale da non continuare ad usare in maniera difforme i fondi per le aree sottoutilizzate, così da orientare la spesa verso le infrastrutture o, comunque, quei servizi che, realmente, producono l'auspicato riequilibrio dei territori, piuttosto che Il FAS, con tutto il rispetto per l'emergenza del problema delle quote latte (che certamente non appartiene al Sud), non può essere utilizzato per queste finalità, ma per permettere di percorrere la tratta ferroviaria Catania-Palermo o quella marittima Messina-Lipari alla stessa velocità con la quale si percorre la tratta ferroviaria Milano-Torino o quella marittima Genova-Isola d'Elba. Se non ci rendiamo conto di questo, non costruiremo mai un Paese che si muove e che cresce alla stessa velocità. Se non ci rendiamo conto di questo, allora non parliamo parliamo, invece, di un Paese schizofrenico. Lo sviluppo armonico dell'Italia ha un costo in termini di solidarietà e di efficienza, ma è un costo che abbatte i costi dello Stato e produce ricchezza. Dunque, è la solidarietà e l'efficienza che dobbiamo realizzare e perseguire con autorevolezza e responsabilità. Concludo chiedendo

sulla riforma federalista nella convinzione che finalmente si sarebbe messo mano a una questione di vitale importanza per il Paese e di grande valore per la politica. Dobbiamo constatare, purtroppo già dall'avvio di tale dibattito, che molte delle aspettative che abbiamo avuto sembrano essere disattese. Il testo, pur migliorabile, ha nei fatti ridotto la capacità di incidenza dello stesso strumento, il quale in più passaggi, talvolta chiaramente e talvolta in modo subdolo, ha ridato fiato a uno dei mali peggiori della nostra politica. Mi riferisco a quel centralismo, a parole aborrito da tutti, ma nei fatti favorito come accade anche in questa riforma sul federalismo. La scorsa settimana è stato ricordato anche in questa sede il novantesimo anniversario dell'appello di Sturzo ai "Liberi e Forti", occasione che forse poteva essere meglioutilizzata, oltre che per le cerimonie di rito, per ritornare con la mente al suo pensiero sull'autonomia, da cui si dipana oggi oggi l'odierno dibattito sul federalismo. Per Sturzo, infatti, l'autonomia degli enti intermedi, la famiglia, gli enti locali, le associazioni culturali e professionali e i sindacati si realizza in uno Stato delle autonomie, cioè che non solo le consente ma si realizza in esse. Il sistema delle autonomie costituisce il complesso di organi adatti alla resistenza contro la potenziale prevaricazione dello Stato ed insieme orientati alla trasformazione della società contro i rischi dell'appiattimento, della conservazione e dell'immobilismo. Le autonomie locali per Sturzo non sono cavalli di Troia da introdurre nella cittadella dello Stato moderno per scardinarlo dall'interno, ma il luogo della partecipazione responsabile delle persone e della vita sociale. Inquesta riforma, purtroppo, si

il feudatario che sta nel vicino territorio; rischieremmo di trovarci con fiato sul collo. Credo che con questa riforma si stia sempre più togliendo spazio di partecipazione ai cittadini e soprattutto alle municipalità - l'aspetto al quale si riferiva Sturzo - per dare più spazio alle Regioni per quale motivo. Èproprio da questa partecipazione responsabile che occorre partire se si vuole che il processo giàmesso in moto non finisca per autocelebrarsi nelle sale delle Aule parlamentari o, peggio ancora, in quelle accademiche.

Vogliamo contribuire ad approvare una legge positiva, purché essa ci aiuti a ristabilire quelle condizioni di parità che si sono invece perse grazie ad un centralismo che, per dirla con le parole di uno della Padania, don Milani, ha commesso la massima delle ingiustizie: trattare allo stesso modo quelli che uguali non sono in questo Paese. Il mio intervento vuole essere un invito ad una più approfondita riflessione su alcuni aspetti che, se non corretti, potrebbero non solo bloccare ogni speranza di sviluppo futuro di larghe aree del Paese, ma anche aggravare questo livello di servizi proprio lì dove c'è più necessità di ridurre le differenze. Il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale si basa sul presupposto che sia possibile innescare, in ambito di governo locale, un circolo virtuoso tra imposizione fiscale e responsabilità politica, perché la politica di trasferimento di fondi dal centro creerebbe un'opacità che impedisce di punire l'amministratore cattivo o inefficiente e di premiare quello capace. Questo discorso, ineccepibile sul piano teorico, non fa i conti con un Paese in cui vi sono ancora Regioni in ritardo di sviluppo, che proprio dal federalismo, da questa legge sul federalismo, attendono la soluzione ad alcuni problemi, che in qualche modo sono atavici (basti solo pensare ai trasporti o alla sanità nel Mezzogiorno). In questo processo, si dovrà tener conto anche della situazione delle cinque Regioni a statuto speciale, i cui statuti sono salvaguardati formalmente dall'articolo 24. Tale salvaguardia, oltre che generica, si rivela nei fatti inapplicabile o comunque priva di effetti, poiché i principi generali che ispirano tutta la riforma non possono non avere riflessi su tutte le Regioni. Infatti, non risulta altrettanto chiaro se con tale disposizione queste Regioni vengano escluse dal meccanismo della perequazione in atto per le Regioni a Statuto ordinario con minore capacità fiscale per abitante. Lo Stato ha il compito di garantire l'imparziale applicazione delle leggi, dei diritti e dei doveri. questo, prima di procedere, occorre si ponga la necessaria attenzione al fatto che se si riducono le tasse, cosa che tutti auspichiamo, o si trasferiscono le stesse entrate agli enti locali per far fronte ai minori trasferimenti dello Stato, per Regioni come la Sicilia, che non godono dei trasferimenti dello stesso Stato, bisogna intervenire con precise entrate sostitutive. Non bastano aleatorie previsioni circa la possibilità che in sede di stesura dei decreti attuativi verranno messe a punto le modalità per arrivare ad una perequazione delle entrate. Si tratta di una previsione troppo generica per poterne tenere conto, che non può che lasciare l'amaro in bocca, soprattutto alla luce delle passate esperienze che ci hanno riguardato come siciliani. Ora, il timore è che se non verrà indicato chiaramente da dove arriveranno i fondi, ci troveremo a dover trovare risorse aggiuntive per continuare ad esercitare le funzioni proprie e quelle delegate negli anni passati dallo Stato ci ritroveremo a dover assumere ulteriori funzioni che comportano costi aggiuntivi, non sapendo da dove e se mai arriveranno i fondi per farvi fronte. Si tratta di milioni di euro, che fino ad oggi, non godendo di trasferimenti da parte dello Stato, la Regione incamerava dalle entrate fiscali che ora il Governo annuncia di voler tagliare. Da domani, se queste entrate cesseranno, con quali fondi la Regione potrà far fronte alle spese per assicurare la parità di trattamenti in materia di sanità, istruzione e assistenza rispetto alle Regioni a Statuto ordinario, o rispetto alle altre Regioni a Statuto speciale, ma con un reddito *pro* *capite* al di sopra della media nazionale? L'alternativa potrebbe essere un aumento delle imposte locali, ipotesi che non è da prendere nemmeno in considerazione, perché risulterebbe altrettanto iniqua, soprattutto per le Regioni più deboli.

Il nostro Paese si fonda sulle differenze territoriali e locali; esse devono essere una risorsa e come tali devono essere valorizzate e sostenute. Il federalismo deve saper rispondere, allo stesso tempo, alle esigenze di specificità e all'interesse all'unità. Torna alla mente

40 minuti; la politica italiana si trova di fronte oggi al disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri il 3 ottobre scorso. Non è il frutto di una novità, ma è la tappa di un percorso avviato con la legge Bassanini del 1998 e, soprattutto, con la legge costituzionale n. 3 del 2001. È un provvedimento che pone all'attenzione di tutti l'attuazione dell'articolo 119 della nostra Carta costituzionale. Si tratta di un disegno di legge che indica all'articolo 2 una serie di aspettative che devono trovare risposta attraverso atti legislativi successivi delegati al Governo. Viene annunciata, cioè, una riforma dello Stato e quindi una nuova fase che attiene ai rapporti tra i cittadini dell'intero Paese. Viviamo, cari colleghi, in un periodo nel quale alcuni vocaboli come «separazione», «divisione», «autosufficienza», «merito», «autonomia» sembrano emergere a dominare uno scenario sempre più illusorio. Che vuol dire federalismo? Quale? Come? Parrebbe essere da alcuni percepito come una forma di riscatto di taluni rispetto ad altri. Emerge, in sottofondo, il rischio che più che di una riforma si tratti di una rivincita di una parte politica che da tempo percorre una strada che fino ad oggi non ha trovato sbocco. noi vogliamo evitare che emerga, in una necessaria e matura riscrittura di alcuni punti cardine utili alla modernizzazione del Paese, quello che definisco l'egoismo dei forti. L'Italia, questo Paese assurto a dimensione unitaria con la gloriosa storia del Risorgimento, questo Paese ritornato libero e democratico con il sacrificio della Resistenza oggi si trova ad affrontare una nuova fase che è matura, che è utile alla costruzione di uno Stato capace di confrontarsi in misura competitiva nel contesto delle nazioni Europee. Occorre però far camminare di pari passo il bisogno di una riforma con l'equilibrio delle distanze, delle differenze che ci sono e che, per certi aspetti, hanno rappresentato fino ad oggi la ricchezza di questo nostro Paese. Ecco allora che il confronto parlamentare deve assicurare il più ampio consenso possibile, considerato il carattere sostanzialmente costituzionale dei provvedimenti relativi alle riforme istituzionali. Occorre, onorevoli colleghi, che la fase attuativa del provvedimento, che consiste nella stesura dei decreti legislativi, con particolare riferimento alle dotazioni di risorse, alla definizione dei LEA e dei LEP, avvenga attraverso un percorso condiviso da Governo, Regioni ed autonomie locali. Il tutto attraverso il coinvolgimento delle Camere e delle Commissioni parlamentari competenti con la previsione di pareri vincolanti sui decreti delegati. Ecco, allora che l'approccio al disegno di legge diviene possibile e doveroso: su tutto deve passare una nuova definizione della responsabilità amministrativa che sappia coniugare i livelli della spesa con l'autonomia dell'entrata. Viene evocato un nuovo concetto, il costo standard*,* un marchingegno che dovrebbe sostituire la spesa storica. Ma quale costo standard? Come? Chi lo definisce? Si dice: rispettando i principi di solidarietà e di coesione, assicurando autonomie di entrate e di spesa, garantendo la loro massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori. Quindi, costi reali di servizi correlati alle funzioni pubbliche attribuite alle autonomie, per meglio utilizzare le risorse del prelievo operato sui contribuenti, purché estese a tutte le funzioni. In ciascuna, infatti, risiede un nucleo di essenzialità, altrimenti sarebbe inutile e dunque semplicemente non andrebbe esercitata. Sui costi standard si gioca quindi la partita più difficile poiché dovranno rappresentare a regime i parametri essenziali per misurare l'efficienza della pubblica amministrazione, sanzionando la eventuale inefficienza. superamento definitivo della finanza derivata. Particolare attenzione merita il fondo perequativo che deve servire a compensare solo quegli enti che non riescono a far fronte alle loro spese con tributi ed entrate proprie e con il gettito della compartecipazione, in quanto il loro livello di capacità fiscale per abitante non lo consente. Ma minore capacità fiscale rispetto a chi? Alla regione più ricca? Da qualche parte politica sembra prevalere il convincimento che la minore disponibilità di risorse per le regioni a minore capacità fiscale, le porterà a far perno sulle loro potenzialità inespresse, avendo la finanza derivata coltivato l'inefficienza della cattiva amministrazione. Il Gruppo dell'Italia dei Valori è per una perequazione verticale: compito esclusivo dello Stato *ex* articolo 117 della Carta costituzionale, comma 2, lettera *e*), è l'istituzione con legge di un fondo perequativo ed il titolare della competenza è il Parlamento della Repubblica. dunque, è uguale a competizione tra territori? Sì, questo sarebbe sicuramente possibile se i competitori alla linea di partenza avessero le stesse potenzialità. Altro punto su cui riflettere è se sia possibile, attraverso l'individuazione di costi standard per tutte le funzioni, riconoscere che vi sono variabili e parametri oggettivi di natura geografica come diceva il mio collega Astore - economica e sociale che lo Stato ha il dovere di considerare, perché se è così, la spesa pubblica per tali funzioni, una volta depurata necessariamente e inderogabilmente dagli sprechi e dalle inefficienze, non può essere ulteriormente comprimibile. Si rende necessario accompagnare il provvedimento con altri urgenti progetti di riforma, come il superamento dell'attuale bicameralismo, attraverso la creazione di una Camera delle autonomie territoriali, con evidente riduzione dei costi della politica ed un più efficace sistema parlamentare in un ordinamento statuale che dopo il 2001 è diventato, come diciamo noi, a regionalismo spinto.

riuscendo ad apportare al disegno di legge alcuni importanti punti, peraltro accolti da parte della maggioranza. Siamo convinti che questa, com'è stato detto da più parti, rappresenti un'occasione storica per la modernizzazione del Paese. È l'Italia che ci sta ascoltando, sono gli italiani. Redistribuire in modo corretto le risorse nel rispetto della piena assunzione della responsabilità politica e amministrativa è la vera sfida che gioca l'avverarsi del federalismo fiscale. Noi crediamo ci siano ancora spazi perché alcuni nostri emendamenti da domattina possano trovare accoglimento. Sì, quindi, ad un federalismo solidale che pone al centro il cittadino, la persona i suoi bisogni e le sue libertà; sì ad un federalismo solidale e responsabile che tenga conto che il percorso da compiere richiede comunque riflessione ed approfondimento. Cara Presidente, cari colleghi del Senato, occorre che l'intero Paese abbia coscienza di questo, di ciò che noi andiamo a proporre. Concludo dicendo no all'egoismo dei forti, sì alla nuova responsabilità. La strada è indicata: tocca alla politica, e solo alla politica, cogliere questo processo di riforma, tenendo conto che l'Italia dei Valori, partito nazionale, farà fino in fondo la propria parte. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo a discutere in questa Assemblea il tema fondamentale del federalismo fiscale, attraverso

della proposta di legge alle Camere approvata dal Consiglio della Regione Lombardia e del disegno di legge n. 1253 del Partito Democratico. Questo provvedimento è scaturito da un clima di fattiva collaborazione tra Governo, maggioranza ed opposizione, e nasce dalla oramai improrogabile esigenza di dare una concreta attuazione alle previsioni costituzionali dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale. La riforma del Titolo V della Costituzione ha posto le premesse per avviare un ampio processo di trasferimento di poteri dal centro alla periferia, incidendo sull'assetto delle competenze e dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali della Repubblica. Tuttavia, perché si realizzi un'effettiva autonomia di Regioni ed enti locali manca un tassello fondamentale: l'attuazione del federalismo fiscale. I ritardi fino ad oggi accumulati nel processo di riforma in senso federale hanno condotto ad una situazione in cui persiste un modello di finanziamento degli enti territoriali "derivato", ossia dipendente dal bilancio statale, anziché autonomo. Ciò ha comportato e comporta ancora gravi disfunzioni nel rapporto tra politica e azione amministrativa e perduranti inefficienze nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Un sistema di finanza derivata, con ripiani a piè di lista alle amministrazioni inefficienti o con criteri basati sulla spesa storica, che ha creato le condizioni per un aumento incontrollato della spesa pubblica, dando la possibilità di scaricare sulla collettività i comportamenti opportunistici di alcuni. Inoltre, tale sistema premia chi più ha creato disavanzi, visto che tanto prima o poi verranno ripianati, e chi più ha speso in passato può continuare a farlo, mentre chi è stato efficiente deve continuare a spendere meno. Questa situazione non è più tollerabile. Si deve abbandonare la logica degli sprechi e l'impostazione centralista ed assistenzialista che ha fatto crescere a dismisura il debito pubblico del nostro Paese. Con questo disegno di legge, finalmente, si va nella direzione del superamento dell'attuale sistema di finanza derivata ispirato al criterio della spesa storica a favore di un moderno assetto di federalismo fiscale, che porti gradualmente al criterio della spesa standardizzata. Sembra un dettaglio tecnico, in realtà è un passaggio importante: il finanziamento per gli enti territoriali dovrà aver riguardo della determinazione dei costi calibrata sulla base di una gestione efficiente ed efficace di una pubblica amministrazione, tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente territoriale ed il numero dei residenti. Viene inoltre previsto un patto di convergenza con cui l'Esecutivo fisserà i parametri che ogni livello di governo dovrà rispettare, sia per quanto riguarda gli equilibri economico-finanziari

e creando un collegamento diretto tra decisioni di spesa e di entrata. Gli amministratori verranno quindi maggiormente responsabilizzati, anche rispetto alla lotta all'evasione e all'elusione, ed i cittadini potranno direttamente valutare l'operato di chi li governa. Dall'attuazione del federalismo fiscale discenderà un nuovo stimolo a comportamenti innovativi e virtuosi da parte di Regioni ed enti locali e più in generale uno stimolo all'efficienza del settore pubblico complessivo. Tenendo presente inoltre che, nel nuovo assetto dei poteri pubblici e delle competenze tra i diversi livelli di governo, le responsabilità legislative ed amministrative degli enti territoriali sono destinate ad ampliarsi in misura significativa. Volumi consistenti di risorse finanziarie dovranno pertanto essere trasferiti dal centro alla periferia a parità di spesa pubblica e pressione fiscale complessiva. Occorre pertanto dare prontamente attuazione alle prescrizioni dell'articolo 119 della Costituzione, assegnando agli enti territoriali le più idonee fonti di finanziamento, adeguate rispetto alle necessità di spesa. È necessario infatti trovare il giusto equilibrio tra autonomia, equità ed efficienza, prevedendo anche per gli enti locali un aumento del grado di autonomia tributaria. Mi preme inoltre sottolineare che, nel testo del provvedimento che stiamo esaminando, si prevede che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non possa produrre aggravi del carico fiscale nei confronti dei cittadini: alla maggiore autonomia impositiva di Regioni ed enti locali corrisponderà una riduzione dell'imposizione statale. L'auspicio è che ogni Regione possa arrivare alla propria autonomia finanziaria, consentendo finalmente ai cittadini di usufruire pienamente dei benefìci e dei servizi derivanti dalle loro imposte. Inoltre, nel testo del disegno di legge delega viene stabilito il principio per cui la perequazione delle differenze delle capacità fiscali sia applicata in modo tale da ridurre le differenze fra i vari territori, ma senza alterare l'ordine delle graduatorie, come avviene già in Germania. Nel nostro Paese attualmente, invece, si evidenzia una stortura negli attuali strumenti di solidarietà interregionale che deve trovare una correzione. Infatti, il sistema vigente risulta totalmente iniquo: per esempio, le Regioni che prima del processo perequativo hanno una capacità fiscale *pro capite* consistente rispetto alla media nazionale, si trovano, dopo il processo di redistribuzione, a scivolare in basso, e viceversa le Regioni "creditrici". Oggi soprattutto i cittadini e le imprese del Nord versano un gettito consistente di tributi che poi però vengono per lo più trasferiti ad altri. Questo meccanismo, se non verrà modificato, rischia di compromettere nel medio periodo la capacità di traino dell'economia del Nord rispetto a quella dell'intero Paese. Con il federalismo fiscale invece si apre una strada nuova, quella che si propone di creare un sistema equo, ma anche semplice, efficace e, soprattutto, trasparente. Costruendo un fisco basato sulla semplicità delle regole si rendono meno gravosi, sia nella percezione che nella realtà, gli oneri per i contribuenti. Si sta andando nella giusta direzione. La nostra gente ci chiede le riforme e per questo ci ha dato la propria fiducia col voto e noi non la deluderemo. Il federalismo è la madre delle riforme ed è alla base di quel cambiamento necessario per dare una reale svolta al nostro Paese. Col muro contro muro oggi non si va da nessuna parte. Ringraziamo tutti quelli che hanno investito nella trattativa dimostrando peraltro come un disegno di legge così complesso sia riuscito ad arrivare in Aula in un tempo così breve, togliendo ogni alibi a chi temeva una perdita di tempo eccessiva con la trattativa tra opposizione e maggioranza.

insieme ai presidenti Azzollini e Vizzini, di presiedere i lavori delle Commissioni riunite e debbo dire che è stato un lavoro serio nel merito, approfondito e con contributi alla luce del sole da parte di tutti, la cui sintesi, fatta dal ministro Calderoli, mi trova totalmente consenziente. È un provvedimento molto importante, strutturale

Come ho già avuto modo di dire in discussione generale presso le Commissioni riunite, la madre di tutti i perché - ripetendo

riportando ai livelli di ogni governo, quanto più possibile, la responsabilità della spesa e dell'entrata.

il bilancio pubblico italiano ha sempre avuto un avanzo corrente di bilancio. Quindi, il deficit per 110 anni è stato legato esclusivamente alla spesa

si è determinato un accentramento delle entrate al 95 per cento allo Stato e un decentramento delle spese al 50 tra Regioni ed enti locali. Si è scollato, cioè, il momento della responsabilità verso i cittadini della raccolta fiscale con il momento della raccolta di consenso presso gli stessi cittadini attraverso la distribuzione di spesa pubblica.

ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della spesa, ridurre gli sprechi responsabilizzando i diversi livelli di Governo e massimizzando il controllo dei cittadini, cioè la democrazia,

ragionevole nel tempo ma definita della pressione fiscale complessiva. Con il federalismo fiscale noi dobbiamo dire ai cittadini a chi debbono pagare le imposte, ma la madre di tutte le domande alla quale dobbiamo rispondere nei confronti dei cittadini è

francamente il rischio forte è che ciascuno corra ad accaparrarsi le entrate e la spesa e nessuno ponga a difesa dei cittadini il vincolo sul totale della pressione fiscale. Non è una questione puramente economica; lo è perché tutti sappiamo che oltre il 40 per cento l'Europa e l'Italia crepano

qualunque forma di governo, di poter leggere liberamente giornali o guardare televisioni: si tratta del patto fondante della democrazia e cioè del crinale tra risorse che restano disponibili nelle tasche delle famiglie e delle imprese e risorse che sono messe a disposizione della comunità attraverso i Governi e i vari livelli di governo.

in primo luogo, applicando il principio di sussidiarietà verticale che non può non partire dai Comuni perché la realtà storica e geografica del nostro Paese e il codice genetico di ciascuno di noi ha nel sangue la comunità comunale. È l'unica realtà storica dalla caduta dell'impero romano fino all'Unità d'Italia. Ecco perché abbiamo impedito che per federalismo si intendesse sostituire lo Stato centrale con 20 staterelli centrali e regionalistici; ecco perché ci sono due fondi di perequazione (uno per le Regioni e uno per gli enti locali), in modo che gli enti locali abbiano certezza e contezza delle risorse che che arrivano direttamente alle comunità locali. In secondo luogo, è evidente - molti colleghi lo hanno già indicato - il percorso parallelo tra risorse e funzioni...

Quindi, lo Statuto delle autonomie e il Titolo V, perché - come è già stato detto - pensare di continuare con 29 materie concorrenti fra Stato e Regioni è irresponsabile. è irresponsabile. Termino, signora Presidente, facendo un piccolo cenno. Ho già detto che, senza un percorso di rientro della pressione fiscale, l'impalcatura rischia di essere pericolosa e di non reggere. Allora mi permetto di segnalare che ho presentato in Aula un emendamento all'articolo 25 in cui, nel totale rispetto dei vincoli finanziari con l'Unione europea in termini di deficit pubblico, chiedo di indicare un percorso morbido, graduale, di sette anni, per tornare al livello di pressione fiscale che il centrodestra aveva ottenuto nel 2006 (il 40,6 per cento) e che il centrosinistra in 18 mesi ha fatto rimbalzare di tre punti, aumentando di tre punti parallelamente la spesa pubblica e non avendo alcun effetto sul deficit. Questo emendamento, che avremo modo di discutere al momento dell'illustrazione, quindi non sfascia i conti pubblici, non ha alcun rischio delle agenzie di *rating*, perché è innestato in una condizione di totale è innestato in una condizione di totale equilibrio finanziario. La scelta politica che deve avvenire in quest'Aula in modo chiaro e trasparente (capisco che la sinistra non la voglia fare, come è già accaduto in Commissione, per codice genetico, perché la sinistra vuole tenersi le mani libere, nel senso che l'equilibrio finanziario del deficit si può ottenere anche aumentando le tasse), la scelta politica che chiedo alla maggioranza e al Governo è di dire con chiarezza che l'equilibrio finanziario, che va rispettato, deve essere ottenuto contenendo le spese correnti e gli sprechi e non caricando di nuovo le tasse su cittadini, famiglie ed imprese. Dichiaro chiusa la discussione generale. Come già annunciato all'Assemblea, le repliche dei relatori e del Governo si svolgeranno nella seduta antimeridiana di domani.